L'ordine del giorno reca: «Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulla composizione del Governo». È in corso la trasmissione diretta televisiva con la RAI che si protrarrà sino alla conclusione dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e riprenderà a partire dalle ore 18.

Signor Presidente, signori senatori, il dibattito di oggi nasce - come sapete - da una sollecitazione del Presidente della Repubblica, al quale rivolgo il mio cordiale saluto. Il Capo dello Stato, con l'autorevolezza che tutti noi gli riconosciamo, ha invitato il Governo a riflettere in Parlamento in merito ai mutamenti intervenuti nella compagine governativa. È un invito opportuno, che accolgo con favore. Sono certo che il Governo uscirà rafforzato da questo passaggio parlamentare. Condivido e rilancio - quindi - l'appello alla responsabilità e alla coesione del presidente Napolitano, convinto che tutte le forze politiche e sociali debbano lavorare nell'esclusivo interesse del Paese, ciascuna interpretando in modo costruttivo il proprio ruolo. Dobbiamo ritrovare l'unità intorno ai valori comuni. Voglio qui innanzitutto ribadire la nostra ferma intenzione di completare il programma di governo per il 2013, arrivando alla scadenza naturale della legislatura. I cittadini potranno giudicare complessivamente il nostro operato attraverso le elezioni politiche generali, come prescrive la Costituzione e come avviene in tutte le democrazie. Se allarghiamo lo sguardo alle grandi Nazioni occidentali, vediamo che né le opposizioni, né i *media*, né l'opinione pubblica reclamano le dimissioni di Presidenti e Capi di Governo in seguito a risultati elettorali di medio termine nelle elezioni locali. La vera anomalia è pretendere la caduta di un Governo democraticamente eletto e, nel nostro caso, legittimato in Parlamento da più voti consecutivi di fiducia. Ecco perché considero le richieste di dimissioni pervenute da esponenti dell'opposizione un mero esercizio di propaganda. Abbiamo il massimo rispetto per il responso delle urne: nessuno tra noi minimizza o finge che non sia successo nulla, ma la richiesta di dimissioni rivolta al Governo è del tutto fuori luogo, tanto più in un momento di oggettiva difficoltà economica per l'Europa intera. Vengo al dunque. Il 14 dicembre 2010 abbiamo scongiurato una manovra di palazzo che avrebbe dato vita ad un Governo contrario al voto popolare del 2008. La maggioranza votata e voluta dagli elettori ha retto quel giorno alla sua prova più difficile, con il supporto di un ulteriore gruppo di parlamentari e restando fedele al mandato degli elettori. La maggioranza e il Governo hanno continuato ad avere piena legittimità sul piano formale e sostanziale. Dopo le dimissioni dei componenti del Governo, a seguito della diaspora che si è verificata nel Popolo della Libertà, abbiamo proceduto al reintegro della compagine di questo Governo che, con la nomina di nove nuovi Sottosegretari, di cui sei eletti sotto il simbolo del Popolo della Libertà, ha raggiunto la quota di 64 componenti, compreso il Presidente del Consiglio. Con le ultime nomine l'attuale Esecutivo resta ancora uno dei meno numerosi rispetto ai Governi che si sono succeduti nella storia recente della Repubblica: ricordo che il II Governo Prodi raggiunse il numero di 103 membri tra Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari. Alcuni dei parlamentari che sono usciti dalla maggioranza, e che erano stati eletti nel Popolo della Libertà grazie a un simbolo su cui era scritto «Berlusconi Presidente», oggi fanno dell'antiberlusconismo la propria bandiera politica. Alcuni di loro avevano fatto del bipolarismo la propria ragione di vita, e si ritrovano ora in un terzo polo che vuole l'esatto contrario. Ma ad essere chiamati trasformisti non sono questi parlamentari che sono usciti dalla maggioranza, ma al contrario quelli che con senso di responsabilità hanno deciso di sostenere il Governo scelto dagli elettori. Io non mi stupisco più di nulla, e so bene che questo è il solito doppiopesismo di un certo modo di fare opposizione, ma tutto questo mi porta a dire che la notizia vera è che l'Italia continua ad essere governata da chi ha vinto le elezioni nel 2008 nonostante il tentativo di realizzare l'esatto contrario. La Costituzione assegna un tempo congruo - cinque anni - nel quale i Governi devono adempiere agli impegni assunti con gli elettori, e noi intendiamo utilizzare proficuamente quello che rimane di questo tempo, nel rispetto del programma votato dagli italiani e nei limiti temporali dettati dalla Costituzione repubblicana. Le elezioni amministrative possono farci riflettere su una più incisiva azione di governo nei prossimi due anni, ma non possono mai influire sulla durata della legislatura che la Costituzione ha previsto e sulla stabilità di un Governo, che trova la sua legittimità nelle elezioni politiche. Chiarito questo punto fondamentale, credo che questo passaggio parlamentare sia utile per ribadire la volontà del Governo e della maggioranza di affrontare con decisione i problemi del Paese. È nell'interesse degli italiani che il Governo completi la legislatura. Potremo in questo modo continuare a mantenere i conti in ordine e completare le riforme strutturali; potremo dare ai mercati quelle garanzie di serietà e di rigore che in questi tre anni ci hanno già consentito di difendere con successo i titoli di Stato; eviteremo certamente di finire come altri Paesi europei che si stanno dissanguando per sopravvivere. Rivendico come un risultato formidabile del nostro Governo il fatto di avere messo al riparo il debito pubblico italiano dagli attacchi speculativi. Sarebbe folle rimettere tutto in discussione e renderci vulnerabili con una crisi al buio proprio ora che dobbiamo agganciare la crescita. Le agenzie di *rating* ci tengono sotto osservazione e le locuste della speculazione aspettano solo l'occasione giusta per colpire le prossime prede che mostrino segni di debolezza. Se il Governo cadesse, immediatamente vedremmo alzare i costi di finanziamento del nostro debito pubblico; dovremmo tagliare risorse alla sanità, alla scuola, alla cultura per pagare i maggiori interessi su BOT e CCT. Sarebbe una sciagura, non per Silvio Berlusconi, non per il Governo, non per la maggioranza: sarebbe una sciagura per l'Italia, per la sua solidità finanziaria, per il suo futuro, per il futuro dei nostri giovani. Questo lo sanno le più alte cariche del Paese, lo sanno i leader politici di ogni schieramento, lo sanno gli analisti politici ed economici, lo sanno i risparmiatori, lo sanno gli imprenditori, lo sanno tutti i cittadini. Il nostro Governo dunque deve continuare a lavorare, perché gli italiani ci hanno scelto e perché abbiamo ben governato, e anche perché - lo dico con chiarezza - non esiste alcuna alternativa a questo Governo e a questa maggioranza. Non intendo polemizzare con le forme e i contenuti espressi dalle altre forze politiche. La democrazia impone il rispetto delle idee altrui anche - anzi soprattutto -quando sono radicalmente differenti dalle proprie. La sinistra può affinare la sua propaganda, può raccogliere qualche voto in più di protesta, può continuare a organizzare il sabotaggio a suon di fischi dei nostri incontri pubblici, può avvantaggiarsi non avendo l'onere di governare il Paese in questi anni turbolenti, ma una cosa è certa: le tre o quattro opposizioni esistenti in Aula e nel Paese sono profondamente divise tra loro e non sono in grado di esprimere un leader o un programma. Non sto dicendo: «Dopo di me verrà il diluvio»: so bene che i cimiteri sono pieni di persone che si ritenevano indispensabili. Mi limito a osservare che l'alleanza tra Popolo della Libertà e Lega, con l'apporto delle forze responsabili del Parlamento, è l'unico assetto politico in grado di garantire la governabilità e l'affidabilità internazionale del Paese. La verità è che le contraddizioni della minoranza sono ben più gravi e radicate dei travagli che la nostra maggioranza ha dovuto subire. può sicuramente dare nei prossimi mesi un importante contributo all'elaborazione di misure e di riforme. Dirò di più, ho sempre auspicato, non solo il sostegno, ma addirittura l'ingresso nella maggioranza, dei settori più moderati dell'opposizione e di tutti coloro che si riconoscono nel Partito popolare europeo, anche se alla mia proposta di alleanza organica e strategica è stato posto un «sì» condizionato alla mia uscita di scena. È del tutto evidente che, sollecitando un suicidio, si esclude in partenza la possibilità di celebrare un matrimonio. Tra i centristi, è prevalso il desiderio di rimanere a giocare di rimessa. Capisco che assumersi la responsabilità di governare è gravoso e che far quadrare i conti dello Stato in un periodo di crisi globale è molto più difficile che fare delle critiche. Ma io non dispero. Sia chiaro, non voglio rimanere per sempre a palazzo Chigi o fare il leader a vita del centrodestra. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Voglio però fortissimamente lasciare all'Italia, come mia eredità politica, un grande partito ispirato al Partito popolare europeo. un partito forte, trasparente, democratico, che sia per il nostro Paese il baluardo primo della democrazia e della libertà. Questa mia apertura non è di oggi, e non è una debolezza, come pure prevedo verrà denunciata a sinistra. Al contrario, è un gesto di stima e di responsabilità: non lascerò nulla di intentato pur di avere una maggioranza e un Governo più forti e autorevoli. Ma per fare cosa? Desidero innanzitutto ricordare i cinque punti qualificanti che il Governo considera strategici per dare attuazione compiuta, da qui al 2013, al programma approvato dagli elettori: il federalismo fiscale, la riforma tributaria, la riforma della giustizia, l'immigrazione e la sicurezza dei cittadini e, da ultimo, ma non per importanza, il piano per il Sud. L'attualità ci ha imposto poi altri temi, dalla vicenda libica alla primavera araba, dal *referendum* fino all'aggravarsi della crisi in Grecia. Quando si guarderà a questi anni di governo con animo meno acceso e mente più serena, non si potrà non riconoscere che siamo riusciti, in una condizione quasi proibitiva, a fare quello che altri Paesi non hanno avuto la capacità o la fortuna di riuscire a fare. Tutti sanno e tutti ci riconoscono che la conduzione della politica economica dell'Esecutivo nel corso della crisi ci ha salvato da una minaccia di *default* finanziario, parola che suona in italiano in modo ancor più sinistro: significa fallimento. Abbiamo trovato nel 2008 l'Italia con un rapporto deficit/PIL superiore a quello dell'area euro. Quel rapporto, da allora, è sempre stato inferiore. Ora è superiore solo a quello della Germania, che non è gravata da nessuna delle pesanti eredità che opprimono il nostro Paese. C'è stato il rischio di essere travolti della crisi e c'è stata la concreta possibilità di subire passivamente tutti gli effetti negativi della speculazione finanziaria internazionale. E invece no. A fronte di scenari catastrofici e nonostante un atteggiamento di diffidenza e mancata collaborazione da parte di molti, non abbiamo solo parato il colpo, ma abbiamo fronteggiato la crisi con autorevolezza e con efficacia, senza ricorrere alle misure che altri Governi sono stati costretti ad assumere, imponendo ai loro cittadini pesanti sacrifici. Alcuni Paesi hanno mandato a casa molti dipendenti pubblici o hanno ridotto fino al 25 per cento i loro stipendi; hanno diminuito gli stanziamenti per la sanità e per gli enti locali; hanno diminuito la cassa integrazione e i contributi ai disoccupati; hanno aumentato l'IVA sino al 25 Il nostro Governo, invece, è riuscito a muoversi addirittura nella direzione opposta, abrogando l'ICI, aumentando di oltre quattro miliardi gli stanziamenti per la sanità e di molto quelli per la cassa integrazione. Il tutto senza aumentare le imposte o introdurne di nuove. Abbiamo fatto tutto questo in presenza di un'economia italiana che ereditava dal passato - e ne è ancora zavorrata - almeno sei gravi handicap strutturali che non siamo ancora riusciti ad eliminare: un debito pubblico che supera di quasi il 20 per cento il prodotto interno annuale e rappresenta il quarto debito pubblico mondiale, senza essere noi la quarta economia del mondo; la quasi totale dipendenza dall'estero in campo energetico, che fa costare l'energia alle nostre famiglie e alle nostre imprese il 40 per cento in più di quello che costa ai francesi; un pesante deficit infrastrutturale, che ostacola la circolazione di merci e di persone, con un costo della nostra logistica del 30 per cento in più rispetto a Paesi come la Germania e come la Francia; un'amministrazione della giustizia civile che ha tempi biblici, fino all'esasperazione; una pubblica amministrazione pletorica e oppressiva nei confronti delle imprese e dei contribuenti; un tasso di evasione fiscale senza uguali in Occidente. dobbiamo avere tutti chiaro che sono proprio tutte queste eredità negative che ci fanno crescere meno della media europea. Nel pieno della crisi mondiale abbiamo poi dovuto affrontare gravi emergenze nazionali: la tragedia del terremoto dell'Aquila, i rifiuti in Campania, gli effetti degli sconvolgimenti africani. A tutte queste emergenze abbiamo dato risposte adeguate e tempestive. Ovviamente non ci siamo occupati solo delle emergenze. In questi anni abbiamo fatto tanto: la riforma delle pensioni, richiesta e apprezzata dall'Europa, ha trasformato il nostro sistema pensionistico in uno dei più stabili dell'Unione europea; la riforma federalista dello Stato, che con l'approvazione dei decreti legislativi sta prendendo corpo e verrà attuata entro la legislatura. Abbiamo realizzato la riforma dell'università e della scuola; abbiamo ridotto drasticamente il numero delle leggi; abbiamo riformato la giustizia civile per renderla più efficiente. Infine abbiamo riordinato e codificato le normative per settori omogenei fino all'emanazione la scorsa settimana del codice antimafia. Abbiamo combattuto la criminalità organizzata e le mafie con risultati mai, mai conseguiti prima: 8.466 presunti mafiosi arrestati; 32 sui 34 latitanti di massima pericolosità, per un totale di 455 latitanti tratti in arresto; 778 operazioni di polizia; 46.569 beni sottratti alla mafia, per un valore complessivo di 21 miliardi e 528 milioni di euro. I progressi nella lotta all'evasione fiscale hanno fatto chiudere il 2010 con oltre 25 miliardi di euro recuperati tra imposte, tasse e contributi evasi. Altri successi: il processo di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, con servizi digitali all'avanguardia in Europa. La diplomazia commerciale che io ho posto al centro del mio impegno in politica estera, ci ha consentito di raggiungere intese economiche per oltre 30 miliardi di euro di commesse a favore delle imprese e dei lavoratori italiani. Voglio poi ricordare che nei mesi più bui della crisi i lavoratori e le aziende non sono mai, mai stati lasciati soli: 37 miliardi di euro di ammortizzatori sociali nel biennio hanno evitato centinaia di migliaia di licenziamenti e garantito il sostegno ai lavoratori, con e senza tutele contrattuali, inclusi i dipendenti di piccole imprese, gli apprendisti, i lavoratori interinali e i collaboratori a progetto. E così abbiamo salvato anche migliaia di aziende. In totale, in questi tre anni di legislatura, abbiamo messo a disposizione del sistema produttivo nuove risorse per quasi 80 miliardi di euro. Queste sono azioni concrete, questi sono fatti, e ringrazio tutti gli italiani che hanno fatto un sacrificio e hanno lavorato duramente per superare il momento più difficile. Signor Presidente, onorevoli senatori, il 6 maggio abbiamo inviato alla Commissione europea il Programma nazionale di riforma e il Programma di stabilità, assumendoci piena responsabilità di fronte ai cittadini e ai partner comunitari. Il giudizio dell'Europa è stato incoraggiante, sia riguardo agli obiettivi per la crescita che al percorso per conseguirli. Il 23 e 24 giugno parteciperò al Consiglio europeo, che dovrà approvare in via definitiva le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea sui nostri Programmi. Subito dopo, approveremo la manovra europea di rigore e sviluppo e vareremo la riforma fiscale, e attueremo il Piano per il Sud. Si tratta dell'implementazione di quanto il Governo ha previsto nel Documento di economia e finanza, approvato dalla Commissione europea e ritenuto adeguato fino al 2012. Prima della pausa estiva adotteremo le misure necessarie a rispettare gli impegni europei, e lo faremo insieme agli altri partner dell'Unione con scelte sostenibili dalla nostra economia. E naturalmente, nella politica di bilancio, il Governo manterrà i suoi impegni, e cioè quelli presi con l'Unione europea, quelli presi con i risparmiatori italiani, con gli investitori internazionali e con tutti quelli che hanno avuto e avranno ragione di dare fiducia all'Italia. Oggi, dunque, il nostro dovere è quello di portare a termine le riforme di tipo strutturale necessarie ad agganciare la crescita. In queste settimane, sui giornali c'è stato un dibattito surreale: si è accreditata l'idea di una spaccatura in seno al Governo. Da una parte, ci sarebbe chi vuole fare una riforma aumentando il deficit; dall'altra ci sarebbe solo il rigore del Ministro dell'economia a difesa dei conti pubblici. Si tratta di una rappresentazione grottesca. Noi siamo tutti convinti - tutti - che non si può aumentare il disavanzo pubblico. Dunque, il Governo non scaricherà sulle generazioni future il costo della crisi economica internazionale, e non farà pagare ai nostri figli le difficoltà del presente. Non lo faremo in nessuno caso e per nessuno motivo. La riforma fiscale non produrrà buchi di bilancio, ma darà vita a un sistema più equo e più benevolo verso chi è in condizioni disagiate. *(Applausi dai Gruppi* chi investe, chi risparmia, chi dichiara il giusto; un sistema più semplice che spazzerà via norme incomprensibili, adempimenti inutili e privilegi corporativi. Il Governo, dunque, presenterà al Parlamento, prima della pausa estiva, la delega per riformare il sistema fiscale. Il Paese ha bisogno di una nuova politica fiscale non soltanto ai fini della crescita economica, ma anche per stabilire un rapporto diverso tra lo Stato e i cittadini. Lo Stato deve fornire dei servizi ai cittadini e alle imprese che è giusto vengano pagati, ma i cittadini devono sentire che ciò che lo Stato chiede loro non è sproporzionato, non è eccessivo rispetto a ciò che dallo Stato ricevono. Come già anticipato dal ministro Tremonti, ridisegneremo l'impianto delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni. Vi saranno meno aliquote (solo tre invece delle cinque attuali), e più basse; un sistema di detrazioni e deduzioni più snello e trasparente, in coerenza con gli obiettivi generali della riforma; una riduzione a cinque del numero delle imposte. Si tratta di un obiettivo non congiunturale, ma strutturale, che rientra negli orientamenti europei da prima della crisi economica, e che in Italia deve portare a riequilibrare il peso delle imposte sui redditi rispetto alle altre imposte, allineandolo progressivamente ai valori europei. Il tutto - voglio sottolinearlo ancora - non in deficit. Non siamo di fronte a una sfida tra coraggio e rigore: si tratta di affrontare, senza demagogia e con senso di responsabilità, una riforma che tutti si aspettano e in cui noi tutti crediamo. La riforma del fisco sarà la seconda fase, il coronamento della politica economica del Governo: prima abbiamo tenuto i conti in ordine, adesso dobbiamo creare le premesse per la crescita. Oltre al decreto sviluppo, il Governo adotterà, anticipandoli in sede di manovra di bilancio, provvedimenti di riforma dell'*export* e del processo civile. Seguirà una serie coerente di altri provvedimenti, per rendere migliore il nostro mercato del lavoro, innalzando la partecipazione delle donne e dei giovani, e per incrementare la produttività del nostro sistema economico. In particolare, un provvedimento, già in avanzata fase di preparazione, riguarderà le costruzioni e le opere pubbliche. Daremo inoltre attuazione concreta al Piano per il Sud,

riuniremo il CIPE ogni mese, con l'obiettivo di deliberare tutte le misure per rendere operativi gli otto interventi prioritari che il Piano stesso prevede. Seguirà la sottoscrizione dei contratti istituzionali di sviluppo con le Regioni e con gli enti interessati per definire responsabilità, tempi e modalità di attuazione. Intendiamo anche apportare un'incisiva modifica al Patto di stabilità interno, così da introdurre meccanismi premiali e meccanismi punitivi Premiali per gli enti locali virtuosi, punitivi per quelli che non lo sono. Solo così potremo superare il cumulo di disposizioni che si che si sono stratificate negli anni e che hanno introdotto correttivi la cui portata complessiva è stata inefficace, se non controproducente. Va poi realizzata la riforma dell'architettura istituzionale. C'è già un'intesa sui princìpi fondamentali riguardanti tre questioni: la riduzione del numero dei parlamentari; il superamento del bicameralismo perfetto, con il Senato federale; infine, il rafforzamento dell'Esecutivo. Prima della pausa estiva, presenteremo il disegno di legge di modifica costituzionale: sarà per il Parlamento un'occasione straordinaria per realizzare una riforma storica. In politica estera abbiamo affrontato vicende epocali, con i rivolgimenti nel Nordafrica, che hanno avuto grande impatto sulle nostre frontiere e sulla geopolitica internazionale. Per quanto riguarda la Libia, sulla base delle decisioni dell'ONU, della NATO e dell'Unione europea, il Parlamento italiano ha autorizzato la nostra partecipazione alla missione internazionale di pace per proteggere la popolazione civile. Ricordiamo che finora, grazie all'azione della NATO, sono state salvate migliaia di vite umane e preservate dalla distruzione intere città. Il Governo italiano si è attivato sin dall'inizio della missione con i partner internazionali per una soluzione politico-diplomatica della crisi, come richiesto dal Parlamento, ottenendo l'accordo del Gruppo internazionale di contatto, che si è riunito qui a Roma lo scorso maggio. Condividiamo le preoccupazioni di quanti temono che siano prolungate le operazioni in Libia, per le quali la NATO ha già indicato il termine di conclusione entro il prossimo mese di settembre. Il Consiglio transitorio di Bengasi, da noi riconosciuto, ha firmato venerdì scorso un accordo con il Governo italiano che consentirà il rimpatrio di cittadini libici e la collaborazione alla prevenzione dei flussi migratori. Infine, si terrà a Roma la Conferenza di riconciliazione libica, dove oltre 200 rappresentanti del popolo libico elaboreranno proposte per il futuro della Libia. In ordine alla diminuzione delle risorse da destinare alle missioni internazionali di pace, il Governo assumerà ogni necessaria decisione dopo l'imminente Consiglio supremo di difesa, presieduto dal Capo dello Stato. In quella sede verrà illustrato un piano di ulteriore contrazione dei costi e una graduale diminuzione dell'entità dei nostri contingenti, sempre in accordo con gli organismi internazionali. Venendo ora agli ultimi accadimenti di politica interna, la scelta degli italiani di abbandonare il nucleare, all'indomani della catastrofe di Fukushima, impone di mettere a punto una nuova strategia energetica nazionale. Il Governo sta lavorando per la diversificazione delle nostre fonti di approvvigionamento al fine di garantirci la sicurezza energetica e di ridurre il costo dell'energia per le famiglie e per le imprese. Dobbiamo anche puntare sulla ricerca e la sperimentazione delle nuove tecnologie, che avranno una quota crescente nella produzione di energia elettrica. Le nuove tecnologie consentiranno di rendere più affidabili e costanti le energie verdi, ovviamente con la dovuta attenzione all'impatto paesaggistico degli impianti di produzione. Signor Presidente, onorevoli senatori, aver salvaguardato il sistema economico e produttivo del Paese è il maggior risultato di questo Governo, il vanto di cui andiamo fieri. Mentre imperversava la crisi, non ci siamo fatti prendere dal panico, abbiamo tenuto la barra dritta e guardato all'interesse dell'Italia. Di questo vorrei ringraziare i colleghi di Governo e tutta la maggioranza, che ha sostenuto il peso di scelte difficili ma necessarie e lungimiranti. voglio ribadire i miei sentimenti di amicizia e di stima nei confronti di Umberto Bossi e di tutti gli amici della Lega. Hanno provato in tutti i modi a dividerci, ma non ci sono riusciti, e non ci riusciranno mai! *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Insieme completeremo anche il federalismo istituzionale, dando ai territori la giusta dose di autonomia decisionale. Questo farà bene al Sud come al Nord e garantirà la crescita di una classe dirigente più responsabile ed efficiente. Ho ascoltato con attenzione le parole del ministro Bossi a Pontida, davanti al suo popolo. Con la Lega c'è un'alleanza leale e solida. Insieme, noi faremo la riforma della Costituzione, la riforma del fisco, la riforma della giustizia, nel totale rispetto del programma votato dagli italiani. Ma non vogliamo fare da soli, chiudendoci nell'autosufficienza della maggioranza: siamo consapevoli di quanto sia importante un largo consenso nelle Aule parlamentari e nel Paese per poter varare le riforme. Per questo saremo interlocutori attenti e rispettosi di ogni vostro contributo. Lavorare insieme sarebbe il modo migliore per rispondere positivamente alle preoccupazioni e all'incoraggiamento del Capo dello Stato, che ci ha richiamati richiamati all'unità nell'interesse dell'Italia; sarebbe anche il modo migliore con il quale tutti noi, che abbiamo l'onore di servire il Paese, potremmo assolvere al nostro compito. È un'ambizione grande, in un tempo di crisi, ma sarebbe anche il modo più efficace per contrastare la crisi. Mi auguro dunque che si possa lavorare tutti insieme affinché l'Italia, al di là della crisi internazionale, possa costruirsi un futuro di maggiore prosperità, di sicuro benessere, di vera giustizia e di vera libertà. Lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo a questo nostro Paese, che noi tutti amiamo. Viva l'Italia. *(Vivi,

Governo. *(Brusìo).* Chi deve lasciare l'Aula, lo faccia con una certa tempestività. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo lavorare, dobbiamo iniziare il dibattito, abbiamo degli orari da rispettare.

dal punto di vista istituzionale e sociale. Mi riferisco alla crisi della giustizia e all'intollerabile situazione delle carceri. Non sono nuove queste nostre sottolineature. Quello che è nuovo è che è forse vero che, da quanto lei ha detto, ne consegue certamente un isolamento politico, ma certo non sociale, che perlomeno 13.000 cittadini italiani in questi due mesi hanno partecipato alle lotte non violente che, in particolare, Marco Pannella porta avanti da due mesi. E io conosco i sorrisi, e conosco le derisioni. Conosco anche un grande protagonista della non violenza, che ha detto: «Prima ci ignorano, poi ci deridono, poi ci combattono, poi vinciamo». Forse, speriamo: perché se vinciamo, forse tornerà a rivivere in questo Paese la speranza della sacralità della legge, sacra perché *erga omnes*, e forse perché tornerà a rivivere il senso dello Stato di diritto, il senso delle istituzioni, il senso dello Stato. Certo, occorre un atto di coraggio e di responsabilità che interrompa una flagrante violenza di Stato. Ho misurato bene le parole, quelle che sto pronunciando. Chi è fuori legge in questo Paese sono lo Stato e le sue istituzioni. E questo non è tollerabile in un regime democratico, perché ne mina alle fondamenta la credibilità verso i cittadini.

era in attesa di una decisione giudiziaria, civile o penale. Se non è un problema sociale questo, allora quale lo è? Da allora la situazione è solo peggiorata. I tribunali penali e civili sono oggi soffocati da 11 milioni di processi pendenti, hanno già prodotto in 10 anni 2 milioni di reati prescritti e continuano a produrre, come una catena di montaggio impazzita, sempre meno sentenze e, al ritmo di quasi 200.000 all'anno, sempre più prescrizioni. Lo chiamiamo Stato di diritto, signor Ministro? Quanto alle carceri, il termine sovraffollamento non rende minimamente la proporzione della catastrofe umanitaria che è in atto negli istituti di pena che molti colleghi di tutti gli schieramenti politici hanno visitato con noi e continuano a visitare, con i detenuti ristretti, davvero, 20 ore al giorno, ammucchiati l'uno accanto all'altro, in celle sporche e degradate, che diventano frigoriferi d'inverno e forni d'estate, nella promiscuità più scriteriata: ci sono detenuti condannati ed in attesa di giudizio, colpevoli in via definitiva ed innocenti fino a prova contraria, prossimi al fine pena o quelli con il fine pena mai. C'è chi è malato e non si può curare, c'è chi è straniero e non viene considerato, chi non ce la fa più e si toglie la vita. Signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, negli ultimi dieci anni nelle carceri italiane si sono suicidati 650 detenuti. A morire in più non sono solo i detenuti: nello stesso periodo si sono tolti la vita anche 87 agenti di polizia penitenziaria. Veda, tutto questo è possibile solo perché avviene nel silenzio e nell'indifferenza del sistema dell'informazione e di quello della politica, con l'eccezione ancora di Radio Radicale, in attesa di sapere se questo Governo deciderà che anche quella voce deve finire di emettere, perché sta a voi decidere, non ad altri. Questo le volevo dire, questo le volevo sottolineare, perché creda: tutte le riforme che lei ha anticipato, se non si basano su un recupero di credibilità, di Stato di diritto, di legalità e di istituzioni, non vivranno neppure lo spazio di un mattino. Signor Presidente del Consiglio, lei è stato un doppio disastro per il Paese e per la Repubblica. Lei ha inquinato la vita politica italiana con il possesso dei suoi mezzi di comunicazione privati e il controllo di quelli pubblici: è sotto gli occhi di tutti la scena miserabile dei suoi esecutori piduisti che dirigono da stanze occulte il servizio pubblico e lo impoveriscono e progettano l'allontanamento degli autori più capaci e più redditizi per la RAI, ma, peggio ancora, lei ha illuso un popolo e tradito tutte le sue promesse. Le sue poche riforme concluse, o sono scatole vuote, come il federalismo (la promessa del decentramento dei Ministeri al Nord mi dà un inconfondibile sapore di farsa), oppure sono danni forse irreparabili, come la distruzione della scuola pubblica, dell'università e della ricerca. Quando questa brutta storia sarà finita, toccherà a noi ricostruire il diritto alla conoscenza e il fascino della ricerca sull'ignoto. Di riforme ne ha concluse così poche che oggi cerca di ingannare ancora gli italiani promettendo loro ancora una volta la realizzazione, in meno di due anni, di tutte quelle che non è riuscito a fare nei dieci anni precedenti, ma di tutte le sue promesse la più fallimentare è lo sviluppo: con lei al Governo, molti, troppi ricchi hanno potuto praticare l'elusione e l'evasione fiscale, mentre il lavoro dipendente sostiene oggi più di qualsiasi altro soggetto sociale il peso della pubblica amministrazione. Con lei al Governo, i giovani hanno scoperto la crescita irresistibile del lavoro precario, a singhiozzo, senza contributi, lavoro nero mal pagato, lavoro gratuito (questo è l'ultimo orizzonte delle scoperte sociali: oggi sono una cifra incalcolabile i giovani dannati al lavoro gratuito). L'unica cosa che ha fatto davvero è aumentare il numero degli irresponsabili nella maggioranza: curioso aumento dell'occupazione! Ma lei finalmente ha perso due volte. Con le amministrative ha voluto forzare un *referendum* su se stesso, e lo ha perso nel modo più plateale. Con leggi mal pensate e mal fatte ha voluto imporre una politica energetica basata sulla ripresa illusoria del nucleare; ha voluto introdurre rapaci privati percettori di tariffe nella gestione dell'acqua, bene comune per eccellenza, e, infine, ha voluto costruirsi l'ultima legge *ad personam* e, per farlo, ha incrinato il principio cardine della Costituzione, l'eguaglianza. Ma, grazie al Cielo, ha perso su tutta la linea! Il voto referendario seppellisce le sue illusioni e, in particolare, pone un ostacolo insormontabile al suo bisogno di autotutela giudiziaria. Il popolo si è svegliato, il Paese le ha tolto la fiducia, la Repubblica saprà impedire il suo irrealizzabile disegno di sedere alla massima carica dello Stato. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, l'addizione di incarichi governativi, all'origine della presente verifica di maggioranza, è occasione di polemica tanto ghiotta e di così facile presa che potrei anche comprendere quelle esigenze spettacolari - chiamiamole così - della sinistra, assai sollecita nell'attribuire scenari di scandalo e malaffare alla parte avversa. Potrei, d'altro canto, ricordare da quale pulpito provengano certe prediche moralizzatrici rammentando, come ha fatto il Presidente del Consiglio, i fasti del caravanserraglio che fu il Governo di Romano Prodi, coi suoi 26 Ministri, 10 Vice Ministri e 66 Sottosegretari, per un totale di 103 membri, non tutti adamantini alla prova dei fatti. Ma anche le argomentazioni della contesa politica che hanno sin qui tenuto banco paiono francamente obsolete, alla luce della grande adunata di Pontida della Lega Nord. Da questo evento, infatti, scaturisce la svolta decisiva che apre nuove prospettive all'azione di governo e che, spero ardentemente, ci lascerà alle spalle gli ossessivi tormentoni, i pantani di parole ed accuse in cui la minoranza sguazza e la maggioranza a volte arranca, distolta dalle cose serie e concrete. Ma le parole di oggi del presidente Berlusconi sono rassicuranti. Quanto alla nomina dei nuovi Sottosegretari, ciò che per noi rileva è l'impegno a condividere il cammino del Governo e a lavorare per portare a compimento il programma premiato dal voto della gente, federalismo *in primis*. Altro non domandiamo loro, nella certezza che sapranno onorare le responsabilità a cui sono chiamati. Ad avanzare pretese di coerenza già ci pensano, mi pare, quei settori che si sono distinti nell'istigare e osannare il voltafaccia di Gianfranco Fini e dei suoi seguaci. Come premesso, ci prefiggiamo di guardare più in là e più in alto della disputa strumentale. È da due decenni che la Lega detta il calendario della vita politica nella Penisola, e certamente non trascurerà l'agenda del Governo che sostiene. Domenica, quando 80.000 padani si sono stretti attorno a Umberto Bossi sul grande prato della città del giuramento, sbugiardando i seminatori di zizzania, è stata acclamata una linea di azione che ora diventa pietra miliare nei rapporti con l'Esecutivo. Crediamo di aver sin qui offerto un contributo determinante ad un Esecutivo a cui, peraltro, vanno riconosciuti i meriti di aver salvato il Paese dalla crisi internazionale senza toccare la sanità, di aver portato a un passo dall'adempimento la riforma federalista, d'aver conseguito nella lotta alle mafie successi mai ottenuti in precedenza. Non possiamo accettare che un Governo di tale statura smarrisca il senso della propria missione riformatrice. Non possiamo più sopportare che non si faccia la nostra parte quando i cittadini sono chiamati ai sacrifici, che ancora non si metta mano con decisione ai costi della politica, a cominciare da quella riduzione dei parlamentari che finalmente possiamo mandare in porto senza indugi nell'ambito della riforma costituzionale di stampo federalista. Non possiamo più permettere che ai costi della politica si aggiungano quelli di improbabili missioni di pace, compiute a suon di bombe sulle città della Libia: una scelta a nostro modo di vedere sbagliata che, oltre a lasciare una tragica scia di morti incolpevoli, scatena esodi incontrollabili e comporta spese belliche ingenti. Ancora, non possiamo tollerare che mentre cifre esorbitanti vengono dissipate nella gestione della cosa pubblica e nelle imprese militari, si impieghi il torchio nei confronti di famiglie e piccole imprese in difficoltà, cioè che i sistemi di riscossione di Equitalia sconfinino in pratiche vessatorie. Queste priorità, contestualmente agli altri punti enunciati a Pontida, ci appaiono irrinunciabili, nella consapevolezza che dalla loro esecuzione, nei tempi rapidi prospettati, dipenderà il nostro rapporto con questo Esecutivo e, ancor più, l'esito stesso dell'attuale esperienza di governo nel giudizio dei cittadini. apre una nuova finestra"). A nome dell'Assemblea, rivolgo un saluto alla delegazione di parlamentari russi, guidata dal vice presidente della Duma, onorevole Alexander Babakov, che sta seguendo i nostri lavori. Benvenuti.

Statuto - «è un movimento politico che, nella consapevolezza dell'appartenenza solidale dell'Italia all'Unione europea, promuove un patto federale tra tutte le Regioni italiane, nello spirito dell'unità nazionale e delle eguali opportunità tra i territori, avviando un nuovo Rinascimento politico italiano. Obiettivo fondamentale del movimento è quello di operare per ridurre le distanze fra le "ricchezze" e le "povertà" sia che esse appartengano alla persona, alla collettività, ai territori».

o al Sud perché non sarà certamente quello che può ridare dignità ai territori più poveri. Semmai potrà essere un'ipotesi di lavoro solo quando e se avremo fatto riforme istituzionali di sostanza, come quelle che noi del Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud abbiamo già presentato: dimezzamento del numero dei deputati, Senato delle autonomie, abolizione graduale delle Province, unione dei Comuni e delle comunità montane sostitutive dei gruppi di piccoli piccoli Comuni, ridisegno del territorio con Regioni per dimensioni più vicine al cittadino. Quando avremo scremato - per così dire - anche i Ministeri, eliminando conflitti di legislazione concorrente, quando li avremo resi più "leggeri", allora potremo riprendere in termini più concreti il dibattito giornalistico di questi giorni. Oggi parliamo di contenuti più attuali, riprendiamo il discorso da quel che avevamo sostenuto il 14 dicembre e che oggi sento il dovere leale di continuare a sostenere *in toto*, a maggior ragione dopo l'esito delle elezioni amministrative, ma soprattutto dopo l'esito referendario. Dobbiamo affrontare rapidamente, con decisione e con saggezza politica, i problemi di democrazia economica, sociale, di rappresentanza, di partecipazione. Dobbiamo prendere coscienza sinceramente e lealmente del fatto che si è rotto il *feeling* con la gente, perché noi siamo una sorta di Parlamento monade, autoreferenziale; ci sentiamo un Parlamento di nominati più che di eletti. Fuori c'è il resto del mondo, la società, il popolo, i tanti giovani e anziani che su un quesito referendario hanno ritrovato la gioia di piangere di emozione soltanto perché hanno partecipato, cioè hanno contribuito a determinare una scelta. A fronte di questi messaggi forti non possiamo rispondere con la sopravvivenza - e sono certa, signor Presidente, che lei non vorrà farlo - ma dobbiamo rispondere con la vita e con la vitalità propria della buona politica, che è tale nella misura in cui sa anche essere umile e sensibile: umile nel riconoscere gli errori e sensibile nel cogliere istanze ed emergenze e trasformarle in azioni positive. la gente ci sta dicendo in tutti i modi, insieme con il Presidente della Repubblica, con i vescovi, che nei lunghi periodi di crisi, quale quello che purtroppo stiamo attraversando, dobbiamo trovare convergenze serie su temi, su temi, pochi, ma seri. Primi fra tutti, Presidente, il pieno riconoscimento dei diritti degli italiani del Sud nel rispetto della Nazione, ed una legge elettorale che consenta la preferenza e riporti il popolo al protagonismo della partecipazione. Nei prossimi giorni daremo vita ad un organismo confederato fra soggetti politici non solo del Sud, ma per il Sud, chiamando a raccolta anche i tanti meridionali sparsi per l'Italia e per il mondo che, con le loro capacità, competenze, professionalità, hanno tanto contribuito a generare ricchezza in altre Regioni. Lo faremo non per chiuderci negli angusti limiti di un soggetto politico connotato da conflittualità con altro soggetto politico dagli interessi territoriali divergenti, ma per aprirci alla costruzione di una grande area di soggetti federati connotata, come invita oggi a fare Veneziani, da un'anima nazionale, mediterranea, che si sappia riconoscere anche nella dottrina sociale della chiesa. Troveremo convergenze - ne siamo certi - su fatti concreti: la riforma del fisco, la riforma elettorale, l'attenzione alle piccole e medie imprese, il quoziente familiare, un federalismo delle pari opportunità per i territori. Un'area che sappia ritrovarsi in valori finalmente e nuovamente riconoscibili e chiari, che voglia agire per eliminare i conflitti che stanno così prepotentemente riaffiorando: le differenze enormi fra ricchi e poveri, fra Nord e Sud, fra datori di lavoro e lavoratori, fra giovani e vecchi, fra uomini e donne, tra precari ed occupati. Un'area che consenta, soprattutto ad alcuni italiani del Paese, di liberarsi dalla schiavitù del bisogno, dalla clientela, dall'arroganza. Se questi sono i presupposti, dobbiamo attrezzarci a dare risposte concrete concrete e realistiche. All'agricoltore del Sud poco interessa che un Ministero stia a Roma o a Bari. Gli interessa di più sapere se il suo Governo saprà fare in modo che Al pensionato a 450 euro al mese dovremo rispondere con un taglio reale e selettivo delle spese, stabilendo un tetto di decenza per alcuni stipendi eccessivi che rappresentano un oltraggio alle tante povertà. Mi sia consentito citare solo un esempio: se per Expo 2015 si consente la deroga al Patto di stabilità per la città e la provincia di Milano, occorre che dal Patto di stabilità siano scorporati i cofinanziamenti comunitari per consentire alle Regioni del Sud di poter utilizzare realmente i fondi che provengono dall'Europa. E prima di pensare a un terzo o a un quarto binario per città del Nord che ne sono già dotate, si pensi alla perequazione infrastrutturale per il Sud, propedeutica, non conseguente, all'applicazione totale del federalismo fiscale, cioè del federalismo solo delle tasse. Probabilmente sarò ancora una volta inserita nella *black list* di coloro che non le dicono che tutto va bene. Sento il dovere civico di dirle, con serietà, con lealtà, con onestà, che molte cose non vanno e che dobbiamo avere la capacità di rinascere, con spirito nuovo, partendo non da fantomatici piani per il Sud, ma dall'attenzione vera per il Sud. Un Sud che è disponibile ad assumersi tutte le sue responsabilità,

Un Governo che voglia partecipare attivamente all'attuazione della strategia 2020 per far uscire dalla condizione di povertà o di esclusione sociale almeno 2 milioni degli attuali 15 milioni di italiani che purtroppo si trovano ancora in una situazione di povertà.

Un emendamento con cui non abbiamo chiesto grandi cose o cose impossibili. Noi siamo assolutamente realisti: abbiamo chiesto, semplicemente, di accelerare l'operatività del Piano per il Sud e di riferire in Parlamento, in tempi brevi, sullo stato di avanzamento dello stesso. dello stesso. Noi meridionali non vogliamo tutto: vogliamo qualche cosa, ma che sia una cosa certa e con tempi altrettanto certi. Le abbiamo chiesto di completare il procedimento di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, anche con il pieno svolgimento della disposizione di delega concernente la perequazione infrastrutturale, prevista nella legge 5 maggio 2009, n. 42. Non pensiamo, signor Presidente, di chiederle molto. Vogliamo continuare ad avere fiducia in lei, purché ci dica con la chiarezza, la lealtà e l'onestà che le sono consuete come stanno le cose: che cosa realmente si può fare e con chi realmente vuole fare queste cose.

ho inteso dare una titolazione a questo mio intervento: «L'esercizio del potere e l'arte del governo». L'esercizio del potere non equivale a governare: l'arte del governare consiste essenzialmente nella lungimiranza, nel vedere più avanti dei governati, studiando e attuando strategie di intervento, anticipando gli eventi. Constatiamo, invece, il fallimento dell'arte del governare a fronte di un esagerato esercizio del potere. L'opposizione - in prima battuta parlo dell'Italia dei Valori - ha svolto e svolge il suo ruolo di critica, di contrasto, di sollecitazione e di proposta. Tantissimi sono i disegni di legge presentati in tutti i settori: dall'economia al lavoro, alla giustizia, alle riforme costituzionali. Questa è l'espressione massima della democrazia; è il presupposto del confronto nell'interesse del Paese. Se non che, noi proponiamo, ma non segue il confronto, in assenza di specifiche proposte nero su bianco del Governo, più incline agli annunci, spesso propagandistici e reiteratamente ripetuti. Il Governo poteva cogliere nelle proposte dell'opposizione il momento del confronto, mentre ha seguito la strada dell'arroganza: ha optato per l'esercizio del potere e l'Italia subisce la parabola del Presidente del Consiglio. La parabola appartiene ai corsi e ai ricorsi storici. Nel suo caso, ci sono state prima l'invidia abbastanza benevola, poi l'adulazione di chi si sentiva coprotagonista, quindi la disistima delle comparse, infine il disprezzo dei delusi. Sino al 2010 lei, signor Presidente del Consiglio, si vantava di un imbarazzante gradimento per la sua persona. Poi, man mano che si staccavano pezzi di sodali e si arruolavano riservisti, si è passati alla tesi di una ritrovata compattezza. Questa progressione evoca il motto «Molti nemici, molto onore». Ora deve correre in tutte le direzioni per mettere toppe alla crisi profonda dell'asserita compattezza: dalla politica estera alla politica del lavoro, alla politica fiscale. Se non che, quando dalle aspettative e speranza dei fatti si passa ai sentimenti e agli stati d'animo delusi, la parabola è irreversibile. Lei parla sempre del suo inguaribile ottimismo: ma quale ottimismo può invocare dai cassaintegrati, dai precari, dai disoccupati, dai pensionati, dai giovani e dalle famiglie? Si è passati dal popolo delle partite IVA al popolo dei pignorati e delle ganasce fiscali. Non si accorge del profondo malessere economico e morale di tanta parte del popolo italiano? Ora propone un programma per il futuro: ma ha provato a fare un onesto consuntivo degli otto anni, sugli ultimi dieci, di di suo governo? Sono tanti, otto anni. Oggi propone toppe e formule, qualche vecchio *slogan*. A noi dell'Italia dei Valori non interessa la persona Silvio Berlusconi, ma preoccupa il fatto che leghi la sua parabola a quella degli italiani. Nel 1945, in pieno crepuscolo, qualcuno pensò all'estrema difesa nel Ridotto della Valtellina aspettando 20.000 fascisti armati che non arrivarono mai. In quella tragica visione crepuscolare si pensava di trasportare le spoglie di Dante Alighieri in Valtellina per dare un segno profondo alla bella morte. Quella storia tragica non le appartiene, anche perché, secondo un proverbio russo, «nessuno mai fu impiccato con i soldi in tasca». Al posto delle spoglie di Dante Alighieri lei vuole portare al Nord qualche ufficio di rappresentanza ministeriale a costo zero; una trombetta di latta per un alticcio Braveheart. Ci eviti il grottesco ed il ridicolo! L'Italia ha bisogno di idee, di progetti e di governo. Lei non è capace di governare e, come tutti gli incapaci, è lesto nel dare sempre la colpa agli altri. Provi invece a chiedere scusa agli italiani. Scopra l'umiltà e ne tragga le conseguenze. Avrà un consenso vastissimo.

Signor Presidente del Consiglio, io non appartengo ad una forza politica che fischia e, in modo particolare, non fischia certamente il Presidente del Consiglio, ancorché personalmente posso non aver condiviso e non condividere l'impostazione che lei ha dato al suo Governo e il suo progetto politico. Quindi, con estrema pacatezza ma con equilibrio, credo di dover dire alcune cose a nome del Partito Repubblicano che qui rappresento, anche in una posizione diversa da quella che ha oggi il nostro attuale segretario, l'onorevole Nucara. A noi repubblicani stanno a cuore due questioni fondamentali, Presidente. La prima è la questione economica, lei l'ha trattata, e certamente ha fatto riferimento alla dimensione non solo nazionale, ma anche a quella internazionale, ai pericoli che il nostro Paese correrebbe qualora si percorresse la strada di una crisi al buio, alla capacità che questo effetto domino possa arrivare anche oltre il Mediterraneo e a Nord del Mediterraneo, e noi di questo siamo ben consapevoli e siamo anche estremamente sensibili Diciamo che sulla politica economica lei sta giocando il futuro del suo Governo e della sua maggioranza, perché sulla politica economica, Presidente, si scommette sul serio,

un Governo in cui, quando si governa, parla una sola persona per tutti, perché c'è un progetto condiviso, un programma condiviso, assunzioni di responsabilità condivise. Il suo Governo non ha quasi mai dato questo esempio. Questo non so se debbo imputarlo al al bipolarismo forzato, che è andato avanti a tutti i costi mettendo insieme il diavolo e l'acqua santa, o se debbo imputarlo imputarlo all'alleanza messa assieme non tanto per seguire un progetto che lei, quando si è affacciato nell'agone politico, ha indicato al Paese facendolo anche sognare

riforme non gliele hanno fatte fare, Presidente, lei deve prenderne atto; deve prenderne atto con forza, con coraggio, richiamando i suoi - non l'opposizione - a questo tipo di responsabilità. Gli impegni con gli elettori si mantengono e soprattutto quegli impegni che avrebbero fatto fare un salto alla nostra economia e consentito al nostro Paese di decollare verso una democrazia più compiuta e verso un impatto con il impatto con il resto del mondo e con l'Europa che oggi non ci avrebbe visto nelle condizioni attuali. Quindi, ben venga puntare sulla crescita,

nella ricerca non soltanto pubblica ma anche pubblico-privata, perché lei sa meglio di me quanto in questo settore siamo indietro. Ricerca di processo e ricerca in senso generale sono due frontiere alle quali dovremmo guardare con maggiore attenzione.

la moralità e il sociale, perché uno sviluppo senza attenzione sociale e senza moralità non è un sviluppo serio, non è uno sviluppo vero. La seconda questione riguarda la legge elettorale.

di cambiare questa legge che non rende giustizia alle aspettative del popolo sovrano, cui lei è sempre molto sensibile, che ha il diritto di scegliersi i propri rappresentanti. Credo che lei intimamente possa convenire con me che non debbano essere i segretari politici a scegliere

Signor Presidente del Consiglio, lei ha avuto un grande merito: senza la sua discesa in campo nel 1994 l'idea liberale sarebbe rimasta marginale nella storia d'Italia. Ha rappresentato un sogno per milioni di italiani, sogno a cui anche io, come tanti altri amici, ho creduto. Lei sa che non ho mai avuto un'ostilità pregiudiziale, né verso la sua persona, che stimo e rispetto, né verso il suo Governo, che ho appoggiato lealmente prima della frattura e con cui mi sono costruttivamente confrontato dopo la frattura con Futuro e Libertà. Ne è una testimonianza il Ministro che le siede accanto, l'onorevole Gelmini, perché la riforma dell'università l'abbiamo fatta insieme. Proprio per questo mi sento legittimato a tenere una posizione che vuole essere chiara e costruttiva. A distanza di 17 anni quel sogno è rimasto sulla carta.

Le sconfitte nei *referendum*, clamorose, con una sua diretta discesa in campo, un suo invito a non andare a votare, a votare, pesano, perché riguardano temi decisivi della politica del suo Governo. In particolare, è decisiva la sconfitta sul legittimo impedimento. Gli italiani hanno scelto di stare dalla parte della legalità.

Quello che lei dice oggi, signor Presidente, in larga misura può essere anche condiviso, ma lo diceva già a settembre. Lo ha detto tante volte in questi anni. Io credo che lei non abbia saputo, voluto o potuto, fare scelte forti e risolutive. Penso, per esempio, alla riforma della giustizia civile a cui lei ha fatto riferimento prima. Una giustizia civile di cui troppo poco si è parlato, affrontata, a mio avviso, in misura del tutto inadeguata nella alla riforma dell'università: una buona riforma che, però, non è stata adeguatamente finanziata. Non vi è stato il coraggio di fare scelte, di trovare risorse adeguate per far decollare veramente l'università italiana. Troppo tempo abbiamo perso a parlare di giustizia penale e nel modo sbagliato e troppo poco invece di quelle grandi riforme che ancora i cittadini italiani attendono; troppo poco tempo per dare risposte concrete ai cittadini italiani. Si è sviluppato anche uno scontro istituzionale che certamente non è solo colpa di questo Governo. Anche alcuni magistrati in passato hanno avuto le loro responsabilità, ma tuttavia questo scontro istituzionale ha fatto male al nostro Paese. L'Italia ha bisogno di una marcia nuova, di un Governo capace di fare grandi riforme, di fare anche quello che non sempre elettoralmente potrebbe essere pagante. La sinistra è ormai, purtroppo, - lo dico con grande franchezza ed amarezza - maggioranza in questo Paese. Io credo che occorra rilanciare il centrodestra. Il PdL si sta sgretolando. Ne prenda atto, signor Presidente del Consiglio: ci vuole una nuova, grande aggregazione dei moderati, un grande progetto politico oltre che un grande progetto di Governo per impedire che questo Paese si avvii verso la stagnazione definitiva ed il centrodestra verso una progressiva dissoluzione. Noi, di Futuro e Libertà, insieme con gli amici del Terzo polo, ci impegniamo per rappresentare seriamente una prospettiva liberale e riformatrice, per dare un contributo costruttivo al rilancio dell'Italia.

Dico subito, per sgombrare il campo da equivoci, che per noi tutti parlamentari e militanti della Lega Nord gli impegni assunti domenica a Pontida da Umberto Bossi sono la nostra bussola, a cui ci atterremo e a cui faremo quotidianamente riferimento anche nelle Aule parlamentari. E di questi impegni programmatici, concreti, chiari e da realizzare entro la fine di quest'anno ne voglio affrontare due in particolare. La Lega Nord, - signor Presidente, lei lo sa - ha sempre perseguito un obiettivo di riforma delle istituzioni per trasformare radicalmente l'assetto di questo Stato; a parole sono tutti a favore di questa trasformazione: da uno Stato centralista ad uno Stato federalista; da uno Stato centralista ed inefficiente, ed inefficiente in quanto centralista, in uno Stato delle autonomie, che serva anche a colmare quella frattura profonda tra Nord e Sud che in 150 anni di storia unitaria non siamo ancora riusciti come Paese a colmare. Ma mentre noi procediamo sulla strada di questa riforma federalista, sono al lavoro le burocrazie parassitarie, statali e parastatali, per difendere i loro privilegi. E quando noi proponiamo un inizio di processo di ristrutturazione territoriale dello Stato federale ed un'organizzazione decentrata dell'amministrazione statale sul modello di ciò che è avvenuto già in altri Stati europei - dove il concetto di grande capitale reticolare diffusa è ormai assodato veniamo letteralmente aggrediti dai falsi federalisti, che scendono in campo a difesa dei loro privilegi centralisti e che resistono con ogni mezzo alla spinta verso la riforma delle nostre istituzioni. Signor Presidente, lei è un uomo del Nord e non è mai stato, e non deve diventare soprattutto ora il paladino del peggiore centralismo statale! Un suo predecessore di centrosinistra nel 1996, 15 anni fa, aveva inserito la proposta della capitale reticolare nel suo programma di Governo, letto alla Camera dei deputati il 31 maggio 1996 in questi termini, che riporto testualmente: "Il Governo intende promuovere il decentramento di strutture o di servizi dall'attuale sede di Roma ad altre città italiane. Ci ispira l'idea di una capitale reticolare che è stata sperimentata con successo in altri Paesi". E aggiungeva Prodi in sede di replica: «Il federalismo è la grandezza di un Paese, un federalismo di cui anche il discorso che abbiamo fatto sulla "Capitale reticolare" è uno degli aspetti fondamentali. Per cui - rispondeva Prodi - alla domanda di Paissan che chiedeva che cosa intendessimo per capitale reticolare, noi rispondiamo che vogliamo cominciare davvero la realizzazione di quello che è negli altri Stati federali, cioè che non solo uffici decentrati ma anche grandi centri decisionali sono distribuiti nel Paese. E cominciamo dalle strutture nuove. Nasceranno le *authority* e queste non potranno nascere a Roma. Saranno l'inizio del discorso del decentramento che comprenderà anche strutture di comando del Paese che ora sono localizzate a Roma e che un Paese federale vede invece vivere in tutto il suo territorio». Signor Presidente, l'Ulivo e Prodi dimostrarono nei fatti che quell'impegno votato dal Parlamento nel 1996 era solo fumo negli occhi, un tentativo di confondere i cittadini del Nord per ottenerne il voto, ma senza voler rispettare gli impegni elettorali. Signor Presidente, lei non commetta lo stesso errore, e soprattutto non ci faccia rimpiangere il pensionato Prodi, che deve rimanere in pensione! La seconda questione che vogliamo sottoporle è legata all'assurdità dei meccanismi del Patto di stabilità, come già lei ha riconosciuto nel suo intervento, che sta strangolando le autonomie locali. Le porto solo un dato, signor Presidente, riferito alla mia esperienza di sindaco di un Comune di 18.000 abitanti: ho un saldo attivo di cassa di otto milioni di euro, ma ho tre milioni di euro di fatture ai fornitori da pagare, e non posso pagarle perché, se lo facessi, salterebbero i meccanismi del Patto di stabilità e subirei le sanzioni draconiane previste dal Patto stesso. Questo sta provocando un disagio enorme ai fornitori del mio Comune e degli altri 8.000 Comuni, che sono piccole e medie imprese, perché la FIAT o la Shell o i grandi gruppi internazionali non sono fornitori dei Comuni. Ho già fatto fallire un'impresa perché non sono in grado di pagare queste fatture, e probabilmente ne falliranno altre. Allora, sblocchiamo, rivediamo questi criteri per i Comuni virtuosi, e consentiamo allo sviluppo economico

nave, abbandoni il ponte di comando, scenda nella sala macchine, rimetta le sue mani nella morchia dei motori e riprenda la guida del suo Governo. Noi saremo al suo fianco. Signor Presidente, esiste un Governo del Paese? Certo, i Governi possono sopravvivere numericamente in Parlamento per qualche tempo, ma se non hanno la vitalità e l'autorevolezza necessarie per l'esercizio della funzione di governo in un tempo di crisi, la loro sorte è segnata. Il suo dimesso discorso di oggi dimostra che non c'è più la vitalità politica per governare.

(per quanto non può essere senza conseguenze essere sconfitti in modo così largo su tre temi strategici per ogni Governo, quali le politiche energetiche, le politiche di liberalizzazione, privatizzazione e salvaguardia dei beni comuni, le politiche per la legalità. Tuttavia, la signora Merkel ha subito una sconfitta forse più grave della sua, ma ha dimostrato di saper reagire cambiando la propria agenda. L'agenda italiana, quella vera e che riguarda tutti, è fatta di due macigni: la scarsa crescita che genera scarso lavoro e una manovra correttiva di 40 miliardi di euro. Qualche giorno fa il Consiglio europeo ha adottato la prima raccomandazione sul nostro

per poter rafforzare significativamente il potenziale di crescita dell'Italia e stimolare la creazione di posti di lavoro». C'è traccia nel dibattito della maggioranza e nel suo stesso discorso della necessità di trovare questa ambizione? Non dire: meglio tirare a campare, se no vincerebbe la sinistra, ci ha detto il ministro Bossi. Ma il Paese non si può permettere di tirare a campare. Ci ha parlato di una delega fiscale, dieci anni dopo la prima e inconcludente delega avuta dal suo Governo, dopo avere raggiunto il record della pressione fiscale dal dopoguerra ad oggi; inoltre, se mai vi fosse questa riforma, avrebbe effetto non prima di due anni. Certo, c'è la grande ricetta dell'unico alleato che le è rimasto: la Lega chiede lo spostamento di qualche decina di ministeriali in Lombardia. Cari colleghi della Lega, a che punto siete!

miliardi non sono, signor Presidente, una tassa imposta dall'Europa, ma il frutto degli errori di conduzione della politica economica del suo Governo; altro che allentare i cordoni della borsa, come si sente dire. La borsa, se c'è, è vuota: a confronto, il mitico tesoretto del compianto ministro Padoa-Schioppa sarebbe la caverna di Alì Babà.

piuttosto che a quella inefficiente: il taglio del 34 per cento degli investimenti, il taglio di 16 miliardi di euro al sistema delle autonomie, presidio della solidarietà sociale del Paese e motore di una committenza pubblica a sostegno del sistema economico. Se la manovra di 40 miliardi si realizzasse, intensificando la ricetta fin qui applicata dal suo Governo, sarebbe una tragedia; può essere invece l'occasione se la si affronta dal lato delle riforme. Lo abbiamo proposto tante volte in questi tre anni: un piano straordinario di abbattimento del debito, un piano industriale della pubblica amministrazione, una redistribuzione del peso fiscale a favore di produzione e lavoro, a danno di rendite ed evasioni. La valorizzazione dei tre grandi *asset* che abbiamo: donne, giovani, imprese innovative. Mi sembra che offriate rassegnazioni invece di riforme, ma il popolo italiano ha deciso di non essere più rassegnato. Direbbe Aldo Moro che è rinato un nuovo senso del dovere, una nuova voglia di riprendere in mano un destino comune, in cui parole come decoro, serietà, solidarietà, pubblico, bene comune tornano a essere parole rispettate. Un Paese così non siete più in grado di rappresentarlo, tantomeno di governarlo.

Signora Presidente, colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio, signori del Governo, l'azione di governo di questa legislatura e lo stesso dibattito di oggi in Aula, che traccia il percorso per i prossimi due anni, sono stati fortemente segnati dalla crisi che ha investito il mondo nel 2008 e dalla sua lunga coda. Valutare questo contesto solo con il metro della strumentalità significherebbe non vedere l'interesse della Nazione. Se invece di questo interesse siamo consapevoli, se esso è più forte della convenienza politica politica momentanea, non ci si può non rendere conto, prima di qualsiasi considerazione, di come la crisi abbia scosso in profondità tutto l'Occidente; di come abbia posto il problema degli squilibri mondiali, della crescita dopata, delle mutate prerogative degli Stati sovrani di fronte alle dinamiche della globalizzazione; di come l'economia abbia finito per investire anche categorie etico-politiche, ponendo la civiltà occidentale di fronte al dilemma di quali siano i principi da salvaguardare rispetto all'effimero di un benessere che si è spinto, a volte, oltre il confine della sostenibilità. Nel nostro Paese la prossima generazione sarà la prima a non avere la certezza di poter vivere meglio della generazione che l'ha preceduta. Ciò impone a tutti di evitare pigrizie, eccessi di strumentalità e anche il rifugio in facili *slogan* ormai fuori dal tempo. Anche noi, signor Presidente, dobbiamo vincere le nostre pigrizie. Continuare, ad esempio, a evocare acriticamente la cosiddetta "rivoluzione liberale", spesso peraltro con un intento polemico, significa riprodurre in maniera stantia formule che oggi, per ragioni storiche e di contesto, hanno perso la carica dirompente che avevano negli anni '90, in un altro mondo. invece bisogno di guardare avanti, non indietro, e di evidenziare oggi quali sono i capisaldi non negoziabili in grado di orientare al fondo l'azione di governo nonostante le contingenze. Per quanto ci riguarda, queste colonne d'Ercole risiedono ad esempio nella garanzia degli equilibri di finanza pubblica, che non è una fissazione di questo o quel Ministro, ma una necessità fortemente avvertita da tutto il Governo e da tutta la maggioranza, non solo in ossequio ai vincoli europei, che passano, ma a presidio di un sistema che sia veramente competitivo e liberale. La politica della spesa in deficit, infatti, prima ancora che miope sotto il profilo dell'efficienza economica, è illiberale ed eticamente ingiusta, perché scarica sulle generazioni future il costo di benefici finanziariamente non sostenibili. Del resto, se avessimo seguito questa linea avremmo esposto il Paese intero alle conseguenze nefaste che altri stanno scontando, perché sanzionati dalla comunità internazionale quando non addirittura minacciati dallo spettro del fallimento. fallimento. È in questi momenti che ci si rende conto di quanto la stabilità sia un bene prezioso. Signor Presidente, un po' come la salute: ci si abitua a darla per scontata, ci si lamenta dei sacrifici che si debbono fare per mantenerla, e la si apprezza o la si rimpiange solo quando viene a mancare. Altro principio irrinunciabile è il binomio costituito dal ragionevole contenimento della spesa pubblica - che concentri l'intervento statale nelle aree di effettivo bisogno, superando l'inefficienza e la crescita autoreferenziale che per decenni hanno caratterizzato le politiche di spesa nel nostro Paese - e dal conseguente alleggerimento della pressione fiscale. Crediamo in un sistema fiscale che oltre ad essere ragionevolmente moderato sia anche coerente con i principi di libertà e responsabilità dei cittadini, che sia a misura della persona e della famiglia, perché se nella nostra società la cellula produttiva del reddito è calibrata sulla famiglia, è inevitabile che, compatibilmente con i conti pubblici e con il contesto internazionale, anche il sistema di imposizione tributaria venga progressivamente adeguato al medesimo parametro di riferimento. Crediamo in un sistema che incentivi la libera intrapresa. Crediamo in un sistema equilibrato che combatta l'evasione anche rendendola poco conveniente, perché se la pressione fiscale e i costi indiretti dell'evasione grosso modo si equivalgono, è evidente che per i cittadini le tasse diventano addirittura invoglianti e bisogna a quel punto pagarle. Crediamo, infine, in un sistema che ponga il mondo giovanile tra le priorità strategiche, perché la vera sfida epocale, signor Presidente, consiste oggi nel rompere quel diaframma che separa la nostra generazione, che si è vista garantire tutele e benefici economici e sociali, dalle generazioni più giovani, che pagano il costo di politiche del lavoro, previdenziali e fiscali pensate decenni fa, quando ad esempio il sistema scolastico e universitario - diciamolo - era pensato più in funzione dei professori che non degli studenti. Insomma, la vera sfida aperta è come tenere insieme stabilità e crescita. E su questa sfida noi ci mettiamo in discussione di fronte al Paese con una proposta chiara, che oggi ci è stata illustrata in questa Aula. Non è una sfida a costo zero, ne siamo perfettamente consapevoli. Ma diciamo che, se siamo pronti a metterci in discussione, c'è una cosa alla quale non siamo disposti a rinunciare, perché è il più grande lascito che questa stagione politica si prefigge di consegnare al Paese. Mi riferisco alla modernizzazione politica e istituzionale che la nostra democrazia, soprattutto grazie alla sua azione, presidente Berlusconi,

l'autentico pericolo è che, con la scusa dei limiti, si finisca con il coltivare disegni di ritorno al passato. A riportare indietro le lancette dell'Italia noi non saremo disponibili. A proposito della legge elettorale, ad esempio, discutiamo di tutto, purché non venga messo in dubbio l'assetto bipolare del sistema e il diritto dei cittadini a scegliersi i Governi. signor Presidente, ha molto a che fare con la stabilità e la crescita. Ha a che fare con la stabilità perché noi non vogliamo tornare alla stagione dei Governi balneari, e non è un caso che l'esecutivo e la maggioranza siano qui oggi, compatti e coesi, a difendere il Governo di legislatura, il Governo che porti a termine il mandato ricevuto dagli elettori. Ha a che fare anche con la crescita, perché non bisognerebbe mai dimenticare che il debito pubblico che grava sulle spalle dell'Italia è figlio innanzitutto dei meccanismi consociativi generati dal proporzionalismo. difendiamo dunque il cammino del nostro sistema politico istituzionale verso la modernità. E su questa base intendiamo ricercare la nuova sintesi possibile tra stabilità e crescita, riempiendo le nostre ricette di un contenuto etico, valorizzando quei beni non effimeri, quelle identità e quelle tradizioni che consentono di sfuggire al falso mito della crescita a ogni costo: anche a costo di scaricare il presente sulle spalle dei nostri figli. Su questo terreno chiamiamo la sinistra chiamiamo la sinistra a una sfida che si fondi sui contenuti e non sui frutti avvelenati di un circuito mediatico giudiziario che si serve di un sistema di intercettazioni che ormai offende non solo la dignità della persona, ma anche

prima o poi. Noi ci auguriamo che abbiate il buon senso di accorgervene prima che sia troppo tardi per tutti e per la nostra democrazia. Noi non sappiamo quale sarà il giudizio che dell'elettorato, alla fine di questa legislatura: legislatura: se ci darà ragione oppure no. Ma se è vero che la politica è durata e continuità, e se è vero che la democrazia rappresentativa implica la sedimentazione di un giudizio, siamo certi di poterci presentare, tra due anni, di fronte ai cittadini a testa alta. Non immuni, certo, da errori e contraddizioni, ma con la coscienza a posto di chi ha lavorato nell'interesse dell'Italia.

la diretta televisiva era stata prevista per le ore 18. Andranno in diretta televisiva, evidentemente, gli interventi a nome dei Gruppi. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18. *(La seduta, sospesa

signor Presidente del Consiglio oggi ha fatto tre affermazioni, tre passaggi che ritengo molto importanti. passaggio è l'esistenza di una maggioranza forte e coesa. esistendo una maggioranza forte e coesa, evidentemente il Governo intende completare il suo lavoro fino alla fine della legislatura. Nel terzo passaggio ha indicato il programma. Questi tre passaggi importanti in linea teorica sono assolutamente condivisibili, anche da parte di una o più opposizioni. Se esiste una maggioranza forte e coesa, intende governare fino alla fine della legislatura su alcuni punti precisi di programma. Lei, signor Presidente del Consiglio, ha elencato questi punti precisi del programma: federalismo fiscale (da completare), riforma fiscale (da fare), riforma della giustizia, controllo dei flussi migratori e programma per il Sud.

del Consiglio, purtroppo - e lei lo sa forse meglio di chiunque altro in quest'Aula e fuori da quest'Aula - devo valutare e ricordare ciò che il Governo ha fatto da settembre ad oggi in merito ad alcuni di quei punti. Circa il federalismo fiscale, è evidente che non si è trattato di spostare sui territori e sui governi territoriali responsabilità e forza, ma di accentrare ancora più le risorse al Governo nazionale, tanto che si sta confondendo il federalismo vero, che dovrebbe spostare i poteri dal centro al territorio, con un dibattito totalmente inutile ed incomprensibile sullo spostamento dei palazzi dei Ministeri centrali,

stretti, non avrei mai voluto commentare in quest'Aula i dati e i numeri relativi a ciò che il Governo ha fatto da settembre ad oggi. Con l'ultima manovra, quella

i restanti 23 miliardi sono stati utilizzati per finanziare 26 miliardi di spesa corrente in più e 3 miliardi di investimenti

che da qui al 2014 nei dati tendenziali le entrate aumenteranno di 93 miliardi di euro.

le entrate da qui al 2014 aumenteranno di 93 miliardi di euro. Di questi 93 miliardi di euro di maggiori tasse che pagheranno gli italiani, 25 miliardi di euro andranno a ridurre il deficit pubblico,

76 miliardi in più di spesa corrente (cifra che comprende certamente i maggiori interessi da pagare da qui al 2014),

tempo di sostenere che esiste la strada per avere rigore e crescita economica...

di ascoltare il Governo per precisare la nuova natura della coalizione politica. E questo è il dibattito che stiamo facendo oggi, perché è cambiata la coalizione di Governo. E penso che questa sarebbe stata una buona occasione per un Governo che avesse avuto la volontà di non ripetere, signor Presidente del Consiglio, gli schemi logori ormai di tutti questi anni: promettere miracoli, realizzare ben poco, compiere errori, dare la colpa a qualcun altro. Questo è stato il meccanismo collaudato

rivoluzione liberale e che oggi, invece, non essendo state messe in pratica, hanno prodotto disaffezione e sfiducia, penso che il Governo abbia dimostrato di non aver colto ciò che è accaduto nel recente voto popolare delle elezioni amministrative

però abbiamo osservato che il bipolarismo all'italiana ha creato più populismo, più estremismo, più conflitti e meno risultati. allora, mi sia consentito dire che l'elogio del bipolarismo che abbiamo ascoltato oggi e la critica ad una rappresentanza proporzionale finiscono nel ridicolo se osserviamo la natura della vostra coalizione.

i Repubblicani, pur gloriosi, il Partito del Sud, la Democrazia Cristiana per le autonomie, i Popolari liberali, la Destra di Storace, la DC dell'onorevole Pizza, il Movimento per l'Italia della Santanchè e i Cristiano-riformisti. Astore)*. E proprio voi venite a parlarci contro lo schema della responsabilità politica di una coalizione coesa alla quale noi vorremmo arrivare?

ma piantiamola con un meccanismo che non ha nessuna possibilità di riuscita». Avrebbe potuto dirci: «Riformiamo la politica». Invece ci proponete di moltiplicare i Ministeri e le loro sedi di rappresentanza - è una vergogna - anziché accorpare e tagliare le Province inutili, anziché concorrere insieme alla riduzione immediata dei costi della politica. Signor Presidente, in conclusione, ci sono due agende possibili davanti a noi, davanti al Parlamento. La prima è quella istituzionale, della convivenza, del dialogo, del rispetto reciproco tra le istituzioni nella politica: quella indicata quotidianamente dal Presidente della Repubblica. Ed è stata presentata nei giorni scorsi un'agenda per l'economia che potrebbe rappresentare un punto di convergenza significativo. Questa non è stata però

i tedeschi sono usciti dalla crisi perché hanno unito le forze e oggi tornano a crescere con la loro economia del 5 per cento perché non hanno fatto tagli

dall'Aula del Senato perché l'agenda del governatore Draghi diventi l'agenda di fine legislatura e affinché l'agenda della convivenza civile proposta dal Capo dello Stato venga assunta veramente da tutti, senza bisogno, presidente Berlusconi, di avversari da additare per prenderli come pretesto dei fallimenti del Governo. Volete una soluzione alla tedesca? L'Italia ne ha bisogno. Volete una soluzione all'italiana? La conosciamo ormai da 17 anni.

Sud)*. Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento con una considerazione più di carattere personale che a nome del Gruppo. a me pare che la pagina di vita parlamentare che, almeno al Senato, si sta oggi chiudendo, trovi - appunto - in questa dinamica parlamentare il suo punto di approdo, mentre la pagina politica resta ancora tutta aperta.

meriti un ulteriore approfondimento, perché altrimenti si rischia la semplificazione e una sorta di lettura autoconsolatoria rispetto a questioni e a problemi di carattere politico che restano tutti aperti. Lei stesso

di rideterminare nuove condizioni di protagonismo e di rappresentanza dentro la vasta area del centrodestra, si è posto l'obiettivo storico, non personale, di consegnare al Paese un grande partito, una grande forza politica, un grande movimento di popolo aperto, dialettico, plurale e capace di rappresentare rappresentare quell'area vasta, quel mondo vasto, quella storia vasta del centrodestra italiano e di determinare quella ricomposizione che è una delle grandi missioni per cui il centrodestra ha senso, storia e prospettiva. Credo che questa sia la cifra culturale, prima ancora che di carattere politico, che deve animare anche la nuova stagione di governo e la nuova stagione politica del centrodestra in Italia:

La frantumazione non è il bipolarismo: il bipolarismo è il tentativo di ricomporre dentro una sintesi di governo la diversità di storie e di forze che si ritrovano intorno a un ruolo e a una missione. Non si tratta dell'utilità marginale: quello è il ricatto bipolare, non la funzione bipolare, ossia la capacità di pensare al bipolarismo secondo il richiamo dello stesso Presidente della Repubblica, quando ci richiama ad una dimensione alta del bipolarismo, che significa democrazia dell'alternanza, competizione leale tra proposte e progetti politici, capacità di recuperare il senso

che non c'è bisogno di meno politica: c'è piuttosto bisogno di recuperare una politica capace di parlare alla gente, al cuore e alla testa delle persone, e di consentire, attraverso nuove forme di aggregazione, la partecipazione e la mobilitazione popolare che dall'emozione dall'emozione si traduca in capacità di cultura di governo, che poi è quello che la politica deve tentare di fare. Ricomposizione delle frantumazioni e delle rotture: la missione che il centrodestra e il Governo devono recuperare è quella di ricomporre la frattura territoriale e generazionale, con una chiarezza di fondo. Lo dico da meridionale orgogliosamente tale. Io rifiuto l'idea del Sud rivendicazionista; io rifiuto l'idea del Sud assistenzialista; io rifiuto l'idea del Sud clientelare; io rifiuto questa cappa di piombo sui meridionali, sulla loro capacità, sulla loro intelligenza *(Applausi dai Gruppi CN-Io Sud e PdL)*, sulla loro fantasia, sulla loro creatività, sulla loro voglia di modernità e di raccogliere la sfida della modernizzazione. Noi non ci tiriamo indietro rispetto alle grandi sfide della modernizzazione e del Chiediamo però che non ci sia neanche l'idea inversa di questo Mezzogiorno demonizzato, di questo Mezzogiorno banalizzato, di questo Mezzogiorno che manca di un racconto, che manca di una storia per colpa dei meridionali, non per colpa della della Lega, di recuperare il racconto meridionale per ritessere dal Sud la trama di una grande idea della modernizzazione italiana attraverso un nuovo modello istituzionale ed un nuovo modello di carattere sociale ricomporre la frantumazione. Noi non chiediamo più risorse, ma chiediamo risorse, qualità e direzione della spesa, che però non può diventare la centralizzazione della spesa, non può diventare una sorta di neostatalismo di ritorno, non può diventare incapacità del dialogo e della collaborazione politica e istituzionale con le Regioni, con le autonomie e con i soggetti sociali. Il Governo recuperi la capacità di direzione, chiami ad un tavolo politico le Regioni meridionali, le forze produttive del Sud e costruisca - quello sì -

un emendamento del Gruppo di Coesione Nazionale nel quale abbiamo detto innanzitutto che il Sud è un interesse nazionale, perché se cresce il Sud cresce l'Italia. Non è un problema soltanto regionale o macroregionale: è un'idea di politica e di geopolitica che guarda al Mediterraneo, alle nuove storie, alla funzione storica che il Mezzogiorno può e deve assolvere nell'interesse dell'Europa, oltre che nell'interesse della comunità nazionale. Pertanto, è troppo piccola la contrapposizione Nord-Sud; non è becera, è stupida, è inutile, sta nella piccola dimensione del provincialismo, non nella grande dimensione dimensione della competizione globale dei sistemi Paese, che mettono a sistema, a regime, a capitale le loro intelligenze, le loro energie, le loro capacità. Noi abbiamo fatto approvare un emendamento che accelerare il Piano per il Sud, riferire in Parlamento del Piano per il Sud e fare un'altra cosa: mettere insieme contemporaneamente il federalismo fiscale con la delega sulla perequazione infrastrutturale, perché il federalismo può tenere insieme questo Paese, può renderlo più competitivo,

e recuperiamo i grandi valori di una tradizione che dentro il centrodestra ha legittimazione e diritto di forza e di protagonismo.

Signor Presidente del Senato, Presidente del Consiglio e membri del Governo, onorevoli colleghi, ancora una volta, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, voglio ringraziare il Presidente della Repubblica che, in assenza di ogni sensibilità del Capo del Governo a chiarire *sua sponte* cosa è successo nella sua maggioranza, lo ha invitato a riferire alle Camere. le ha chiesto formalmente di investire il Parlamento delle novità intervenute nella maggioranza che sostiene il Governo, rilevando che sono entrati a far parte dello stesso esponenti di Gruppi parlamentari diversi rispetto alle componenti della coalizione che si è presentata alle elezioni politiche del 2008. Un vero e proprio ribaltone, degno del peggior teatrino della politica, che lei, sempre e solo a parole, Presidente del Consiglio, ha finto in questi anni di combattere. A dir la verità, ero sinceramente curioso di sapere cosa ci avrebbe raccontato oggi, come avrebbe giustificato l'improvvisa e assoluta necessità di coinvolgere nell'azione di governo nuove figure, e come avrebbe spiegato il contratto di mera convenienza - perché di questo si è trattato - stipulato con i vari disponibili a tutto, raccattati alla fine dell'autunno del 2010 e ricompensati con un posto, dato o promesso, di Sottosegretario, per la fiducia del 14 dicembre Ma poi, riflettendo meglio, la mia curiosità si è trasformata nella certezza che la sua presenza oggi e qui, in questa Aula, non abbia alcun senso. La vera anomalia è che lei ancora non si sia dimesso, ma non per quanto successo alle elezioni amministrative o al *referendum*, bensì per il fallimento totale delle politiche del suo Governo e il logoramento vieppiù visibile della sua *leadership*. In verità, avrebbe dovuto farlo da tempo. Avrebbe dovuto prendere atto che gli italiani non hanno più fiducia in lei. E in lei non hanno più fiducia neppure molti dei suoi stessi parlamentari, che ormai provano a riposizionarsi per sopravvivere al crollo di un sistema. Gli italiani glielo hanno gridato in faccia, Presidente, in modo forte e chiaro con il voto delle amministrative, vinte dal centrosinistra, con programmi veri e credibili e candidati forti e graditi alle loro comunità; amministrative vinte da noi e perse da lei, che improvvidamente le ha trasformate in una ordalia sulla sua persona. Il suo *appeal* è venuto meno, la sua capacità di imbonitore si è disintegrata e questo per le difficoltà in cui versa il Paese. La gran parte dei cittadini deve combattere le negatività di ogni giorno: disoccupazione, salari sempre più miseri, precariato, cattivo funzionamento dei servizi pubblici, alta pressione fiscale, povertà sempre più diffusa, corruzione dilagante, consorterie di ogni teppa. E se non bastasse, i *referendum*, che il mio partito, l'Italia dei Valori, con orgoglio ha promosso e ha generosamente messo nelle mani degli elettori come patrimonio comune, hanno ribadito la sua *défaillance* perpetua. Le sue politiche sono state strabattute: niente nucleare, niente più leggi *ad personam*, né oggi né domani, per affrancarla dai processi, niente acqua privatizzata. Per questo, presidente Berlusconi, la sua presenza qui rappresenta un nonsenso, mentre, se avesse rassegnato le dimissioni, non avremmo dovuto neppure ascoltarla raccontare in verosimili storie di come e perché ha dovuto indicare ben nove Sottosegretari che, fino a prova contraria, non risultano aver ricevuto alcuna delega specifica. Costi, Presidente, costi della politica: quelli che i suoi alleati leghisti dicono a parole di voler combattere, pronti poi a trasferire i Ministeri in giro per il Paese, evidentemente non pensando ad un aumento della spesa. Le sue dichiarazioni le riteniamo, come Italia dei Valori, sciatte, inconcludenti, inutili, senza speranza per il Paese; in una parola, ripetitive di quanto detto negli ultimi 17 anni. Presidente Berlusconi, lei sta tenendo in vita il Governo solo grazie a riti *voodoo*. Va avanti a forza di trucchi come la compravendita parlamentare per ottenere una striminzita maggioranza, l'approvazione di leggi canaglia per i suoi guai giudiziari, il sostegno osceno a *lobby* e cricche. Mi perdoni, ma le sue arti da prestigiatore hanno ridotto la maggioranza che governa il Paese a un fantasma politicamente senza vita. Siamo di fronte al peggior ammasso - e non lo ricordo solo io - di partiti e partitelli della storia, gente che entra e che esce, tutto e il contrario di tutto. Non c'è chiarezza né trasparenza di linea politica perché i suoi veri ispiratori sono il sottobosco del potere e i bassifondi del clientelismo. Lei ha portato in Parlamento - e se si considera la sua storia personale non ci meravigliamo -rappresentanti della P2, della P3, della P4, il cui metodo di lavoro è di imporre la volontà della cricca ai centri decisionali del Paese con la logica della affiliazione e del ricatto, dello scambio di favori e del dossieraggio. Ma di quale mutamento della maggioranza ci è venuto a parlare? Forse un mutamento genetico c'è stato perché, anziché davanti ad una maggioranza, siamo di fronte ad un mostro politico. Ecco perché, Presidente Berlusconi, la sua presenza in quest'Aula non ha più senso. Lei annuncia un'improbabile riforma fiscale, pur sapendo che dovrà essere varata una manovra da 45 miliardi di euro, che ricadranno sicuramente sulle fasce sociali più deboli. Veda, Presidente, è dal 1994 che ripete le stesse cose, ed è strano che un uomo che sui media ha creato la sua fortuna non si accorga non si accorga che va ripetendo cose vecchie e stantie, senza convinzione e senza passione, e parlando a sale tristemente vuote, dove nessuno l'ascolta. Sì, ormai parla da solo, a se stesso, e probabilmente non riesce neppure a convincersi! Ecco perché la sua presenza, qui ed oggi, non ha più senso. Presidente del Consiglio, non so se lei se ne è accorto,

che si muove in senso opposto al suo stanco e flebile vivacchiare nelle chiuse stanze di Palazzo Chigi. C'è partecipazione dei giovani, che tornano ad essere finalmente protagonisti. Di che si tratta? Lei sorride, Presidente. Forse è una parola che non conosce. E' la democrazia, che grava sulle sue spalle come un macigno, e per quanti sforzi faccia non riuscirà a liberarsene. E' la democrazia quella effervescenza che si respira nelle piazze, tra la gente, nei movimenti della società, che chiedono a gran voce un cambiamento: e cambiamento sarà. sarà. Presidente, stiamo per entrare in una fase nuova della politica. Non me ne voglia, ma lei non ne farà parte. Non lo stabilisco io, ma la ineluttabilità storica delle dinamiche sociali. Lei rappresenta il passato; il berlusconismo è un dinosauro della politica ormai avviato all'estinzione. Il Paese deve fare a meno delle contrapposizioni, e per farne a meno deve necessariamente partire dalla sua salita al Colle per rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.

Allora, fresco di un importante successo elettorale, ci spiegò che, finalmente libero da ogni condizionamento della vecchia politica, avrebbe modernizzato l'Italia, trasformando in realtà le tante promesse fatte in campagna elettorale. A distanza di tre anni ci ritroviamo in quest'Aula a fare un bilancio negativo della sua attività e a constatare che lei presiede un Governo immobile, prigioniero delle sue beghe interne; un Governo che, a differenza di quanto lei dice, non ha mai voluto confrontarsi con le opposizioni, e meno che mai con la nostra, quella del Terzo polo, che si è sempre resa disponibile ad un confronto sereno sul merito dei problemi. A tale riguardo, le vorrei dire, signor Presidente, che, da che mondo è mondo, chi è all'opposizione e si acconcia con il potere è un trasformista, e non chi, a testa alta, dissente e si dimette. Quanto a noi centristi che, com'è noto, lei ha sempre intimamente amato, vorremo ricordarle che siamo sempre stati coerenti con i nostri valori e programmi e stiamo dove ci hanno collocato gli elettori nell'ultima competizione elettorale, perché, a differenza di altri, noi non siamo in vendita e il confronto lo facciamo nella sede naturale della sovranità popolare, che è il Parlamento, e non a Palazzo Grazioli. Lei, signor Presidente, e la sua maggioranza a trazione leghista avete preferito al confronto alla luce del sole l'antica quanto detestabile pratica del trasformismo parlamentare, mercanteggiando con singoli deputati e senatori per far nascere l'Esecutivo che passerà alla storia con il nome di Bossi-Scilipoti: una formula che è la plastica rappresentazione di quel teatrino della politica che da decenni lei e il leader leghista a parole dite di voler contrastare, un teatrino che domenica a Pontida ha dato il meglio di sé. Oggi, proprio per la sostanziale mutazione del Governo, perché pezzi importanti della sua maggioranza sono passati all'opposizione e pezzi d'opposizione sono entrati in maggioranza o, peggio ancora, nell'Esecutivo in violazione di ogni elementare regola di trasparenza e lealtà nei confronti degli elettori, le è stato chiesto di riferire in Parlamento, in questa sede le diciamo con chiarezza e serenità che non è scimmiottando la prima Repubblica che ve la caverete, né riesumare vecchi *slogan* e fare il *restyling* della vostra propaganda fallimentare vi servirà ad uscire dalla profonda ed irreversibile crisi politica in cui siete caduti. Questo Governo, purtroppo, non ha la forza di affrontare i problemi dell'Italia e non gode più, peraltro, di un ampio consenso popolare, come dimostrano i risultati delle elezioni amministrative e dei *referendum*. Avete la maggioranza in Parlamento, ma non nel Paese e continuate con questa spocchia sinceramente incomprensibile. Il Paese è stanco di promesse e di annunci ed è appesantito da una crisi economica che ha fiaccato le famiglie e le imprese. La nostra economia non cresce e ciò nonostante bisogna fare un'altra manovra economica che si attesta sui 40 miliardi di euro per tenere sotto controllo i conti pubblici. In una fase di recessione, questa manovra, che tentate disperatamente di nascondere all'opinione pubblica, sarà prevalentemente a carico dei soggetti più deboli, come le famiglie, sia quelle numerose che quelle monoreddito alle quali avete promesso, mentendo, il quoziente familiare, quando ora si ritrovano a pagare un progressivo aumento delle tariffe dei servizi pubblici e dei prezzi dei beni di prima necessità. invece, essere grati alle famiglie italiane per aver garantito con i propri risparmi la nostra credibilità in sede europea supplendo anche alle carenze della politica del Governo. Dovremmo essere loro grati anche perché le nostre famiglie, tanto al Nord quanto al Sud, stanno mantenendo i giovani disoccupati e i giovani precari - gli stessi che voi insultate - evitando l'acuirsi di una crisi sociale e generazionale senza precedenti nel nostro Paese. Signor Presidente, è proprio sui contenuti che non ci intendiamo: ogni volta che il Governo è in difficoltà evocate la riduzione delle tasse, e poi non la fate, perché non si può fare. I tagli fatti e quelli da fare servono infatti a mantenere gli impegni in Europa e ad evitare di fare la fine della Grecia e non si possono impegnare, quindi, per ridurre le tasse, né potete spacciare per riforma una mera operazione di *restyling* del sistema che non tocca in alcun modo il livello della pressione fiscale. A ciò si aggiunga che con la manovra dell'agosto scorso avete tagliato circa 10 miliardi di euro a Regioni ed enti locali e che con i decreti attuativi del federalismo fiscale avete dato in cambio alle Regioni e al sistema delle autonomie la possibilità di aumentare le tasse. È, pertanto, ovvio che Comuni, Province e Regioni aumentino progressivamente le tasse per coprire i costi dei servizi e che il conto siano costretti a pagarlo, ancora una volta, le famiglie e i ceti più deboli. Avete evitato di mettere direttamente le mani nelle tasche degli italiani, costringendo gli enti locali a farlo al vostro posto. Come se tutto ciò non bastasse, in questa difficile condizione economica interna ed internazionale vi avvitate in discussioni di lana caprina disquisendo se al Nord debbano andare i Ministeri o loro sedi di rappresentanza, confidando ancora una volta nell'indulgenza degli italiani. Noi abbiamo pudore e a questo finto dibattito non partecipiamo; diciamo solo che con il vero federalismo i Ministeri si chiudono e non si trasferiscono, né si aprono miniambasciate italiane in Padania, buone solo a sperperare soldi pubblici. *(Commenti dal Gruppo LNP).* Voi, i Ministri e i Sottosegretari li avete aumentati. Spendete e spandete in danno dei contribuenti, come avete fatto con le Province, che avevate promesso di sopprimere e che tenete lì perché avete i presidenti leghisti attaccati alla «cadrega», come avete fatto per la riduzione del numero dei parlamentari, che tirate fuori quando la gente protesta e poi dimenticate quando non sentite più il fiato sul collo dell'opinione pubblica. A proposito, signor Presidente, le do una notizia: la riforma epocale della giustizia e dell'architettura istituzionale non la potete fare perché, come è noto, mancano grosso modo diciotto mesi alla fine della legislatura, e diciotto mesi sono pochi per cambiare la Costituzione. Per non parlare delle mancate promesse sulla sicurezza e sull'immigrazione clandestina: le ronde sono state un *flop*, i clandestini condannati per gravi reati sono ancora lì in carcere e non li avete espulsi, come non avete espulso gli irregolari perché con il taglio dei fondi alle forze di polizia avete reso impossibile l'accompagnamento alla frontiera. I militari in strada sono stati un altro costosissimo *flop*. Per nascondere il vostro fallimento sul fronte della sicurezza dovete trovare l'ennesimo capro espiatorio e dite che la colpa è del conflitto libico, assecondando irresponsabilmente le sparate di Pontida sul ritiro degli italiani dalle missioni internazionali di pace. Sappiamo tutti bene che dobbiamo stare in Libia finché non si caccia Gheddafi, e sappiamo tutti bene che gli sbarchi non iniziano e non finiscono con la nostra uscita dalla missione in Libia, perché sono frutto di un cambio epocale nella società africana che ha visto crollare regimi che governavano quei Paesi da trent'anni. Tutto ciò è chiaro: basti pensare ai 25.000 tunisini in fuga dalla guerra civile che sono venuti in Italia e che nulla hanno a che vedere con la Libia. Signor Presidente, la verità è che la politica estera non si può fare con lingua biforcuta. Gli impegni internazionali dell'Italia non possono essere merce di scambio politico, né si può dire una cosa a Bossi e l'esatto opposto ad Obama per tirare a campare. All'estero dubitano di noi, mentre in Italia non vi crede più nessuno, a cominciare dal Mezzogiorno, che avete abbandonato sacrificandolo sull'altare dell'accordo politico con la Lega. Niente fondi per il sostegno alle aree depresse, niente infrastrutture, nessun intervento concreto di alcun genere e tipo. Il tentativo l'altro giorno alla Camera di buttare fuori dalle graduatorie del Nord gli insegnanti meridionali è a dir poco vergognoso. Assistiamo impotenti ad un continuo, progressivo e strutturale indebolimento delle politiche per la crescita del Sud. Attenzione, non stiamo parlando di soldi per fare assistenza, stiamo parlando di risorse indispensabili per rendere il Mezzogiorno soggetto attivo e competitivo nel mercato interno e internazionale. Continuiamo ad ascoltare solo chiacchiere e promesse, a partire dalla Banca del Sud, di cui non si ha più traccia, e dal Ponte sullo Stretto, che, visto come è combinata ancora oggi la Salerno-Reggio Calabria, non vedrà mai la luce. Signor Presidente, le sue comunicazioni non ci meravigliano affatto: sono l'ennesimo, edulcorato bollettino di guerra, funzionale a tenere in piedi una maggioranza che non è più nella condizione di governare il Paese. Lei e l'onorevole Bossi prendete tempo e vivacchiate nel disperato tentativo di sopravvivere al fallimento della vostra alleanza e del vostro Governo: sembrate Totò e Peppino a Milano. Siete ed apparite spaesati, parlate un linguaggio ormai incomprensibile alla società italiana, per esorcizzare la fine di una stagione politica che, purtroppo per voi, si è conclusa nel cuore degli italiani già da tempo. L'Italia ha bisogno di un Governo stabile ed efficiente, e non della controfigura di un potere, il vostro, privo ormai di credibilità e autorevolezza. al Presidente del Consiglio che il Movimento per le Autonomie non avrebbe più votato la fiducia al suo Governo, sfuggii da qualsiasi argomento che fosse collocabile in quella cronaca politica che che sforava nel *gossip* e nella cronaca giudiziaria, e rimasi legato rigidamente alla condizione di fondo che aveva determinato l'accordo politico tra il Movimento per le Autonomie, la sua coalizione e il suo Esecutivo: le politiche per il Mezzogiorno. Sento con piacere che alcuni miei colleghi hanno già evocato il problema, e devo dire che nell'intervento del collega Viespoli c'è il fallimento del suo Governo. Viespoli è stato costretto ad un intervento di grande passione, richiamandola ad una nuova prospettiva, perché, nei fatti, questo Governo in tre anni non ha operato per nulla. E quando a dicembre rompemmo il patto di solidarietà che ci legava al suo Esecutivo, affermammo ragioni precise, facemmo i conti, conti, costringemmo il Ministro dell'economia a dare conto della piena inattuazione del punto 5 del programma di Governo che - ricordo - fu scritto insieme, fu scritto insieme, alla vigilia di quella campagna elettorale che poi la vide prevalere con grande successo nel Mezzogiorno. Questo è accaduto perché il suo Esecutivo è sbilanciato culturalmente e politicamente. Su di esso grava l'ipoteca della Lega Nord, un'ipoteca che oggi diventa ancora più pesante quanto più debole è la sua azione politica, dal momento che le ultime vicende elettorali la interrogano in modo significativo sulla prospettiva di questo Esecutivo. Come gli animali feriti, la Lega oggi è più pericolosa per il suo Governo, signor Presidente, e lo è per il Paese e per la sua coesione nazionale. del Consiglio, lei ogni tanto evoca De Gasperi, ma consiglierei al dottor Letta, che De Gasperi l'ha conosciuto davvero, di sconsigliarle questo paragone, non solo per ragioni di etica pubblica e privata, ma per ragioni di cultura politica. De Gasperi, che definiva questo Paese stretto e molto lungo, si fece carico di un'azione finalizzata a tentare di cucire la frattura drammatica che sta sopra il Garigliano e che scandisce il divario tra due aree aree profondamente diverse. Qualche settimana fa, quando l'ISTAT ha reso noti i dati sullo sviluppo, dichiarando che il Nord aveva indici di crescita in linea con il *trend* europeo, il Centro stentava ma avanzava, e il Sud era fermo, rappresentava certamente una condizione oggettiva differenziata legata al reddito, alle infrastrutture, alla qualità dei servizi e al sistema delle imprese, ma enunciava anche il manifesto chiaro degli effetti della vostra azione: tre anni di azione politica di questo Governo sono stati caratterizzati dal trasferimento di ingenti risorse destinate alle politiche di coesione per garantire i livelli di benessere e di tenuta del sistema economico e delle famiglie del Nord.

scontano ritardi assolutamente sovrapponibili a quelli delle Regioni e delle autonomie meridionali. Il fatto è che in termini di sistema Paese non si riesce a concepire davvero, anche per la cultura politica che ispira questo Governo, uno sforzo di recupero e di coesione nazionale. Signor Presidente, lei non può evocare oggi una situazione di riconciliazione nazionale e di coesione nazionale, perché lei non è uomo della riconciliazione, lei non può fare appello ai moderati, perché lei non è un moderato. Lei è l'uomo che si è nutrito di questo bipolarismo muscolare e quando si richiama al popolarismo ...Quella è una cultura diversa. Lei lo avverte solo come la propria parte da scagliare contro l'altra parte, che per lei sono avversari.

il messaggio che hanno voluto darci i nostri elettori alle ultime elezioni amministrative è stato molto chiaro: un messaggio che la Lega non ha voluto in nessun modo sottovalutare. Altrettanto chiaro è stato il messaggio che il grande raduno di Pontida ha dato al Governo e alla maggioranza domenica scorsa.

al nostro territorio. È questo che chiedono i cittadini al Nord, in Padania, e, ne sono convinto, anche nel resto del Paese. Risposte che noi vogliamo dare da subito. Ci vuole dunque un'accelerazione forte e radicale nell'azione della maggioranza. Tanto per essere chiari, e mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza, non è pensabile rimanere al Governo e vivere alla giornata. Su questo, penso che siamo tutti d'accordo. Cosa vogliamo come Lega? Fatti, leggi e riforme in tempi certi. Cosa chiediamo? Una serie di misure concrete che puntino a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e a rendere più moderna, una volta per tutte, la macchina farraginosa di questo Stato. Chiediamo l'approvazione di misure per la riduzione delle bollette energetiche. Chiediamo interventi a sostegno del settore agricolo e degli allevatori. Chiediamo la riforma del patto di stabilità a favore dei comuni virtuosi. Chiediamo che nella prossima manovra fiscale non ci siano tagli agli enti locali e norme penalizzanti per gli artigiani, per i commercianti e per i piccoli imprenditori, che in questo momento sono in ginocchio a causa della crisi economica. Chiediamo di smetterla con le vessazioni di Equitalia: come è già stato detto in quest'Aula da altri colleghi della Lega, non si può pignorare un'automobile o una casa a chi, in un momento di crisi, non riesce a pagare una multa. Siamo consapevoli della crisi economica che stiamo vivendo, ma siamo convinti anche che sia necessaria una seria riforma fiscale a sostegno del settore produttivo e delle famiglie. Chiediamo l'approvazione di una riforma costituzionale, con la riduzione del numero dei parlamentari, con la fine del bicameralismo perfetto e con l'istituzione di un Senato federale. Chiediamo un taglio serio ai costi della politica.

costano. Ci vogliono i soldi per fare le guerre e, in questo momento, soldi non ce ne sono. Ho illustrato diverse delle nostre richieste; sono richieste chiare. Non chiediamo nulla d'impossibile, e siamo convinti che in questo modo, in pochi mesi, riusciremo a dare quella svolta all'azione di governo che con forza ci chiedono i cittadini. In questa legislatura, come maggioranza - è giusto ricordarlo, e per questo voglio ringraziare anche i colleghi del Popolo della Libertà - abbiamo già fatto vedere che, se vogliamo, i risultati importanti si possono ottenere. le spese dello Stato tagliando sprechi ed enti inutili. Abbiamo investito miliardi di euro negli ammortizzatori sociali, salvando migliaia e migliaia di posti di lavoro. di lavoro. Abbiamo approvato il federalismo fiscale, che fra poco entrerà in vigore, e abbiamo contrastato le mafie e la criminalità come mai nessuno in passato. Sono risultati che la sinistra al governo non è mai stata in grado di ottenere. Bisogna dunque solo crederci e lavorare tutti insieme con grande determinazione. E per questo voglio ringraziare i Ministri della Lega Nord, perché si sono già mossi, all'interno del Governo, facendo vedere la giusta reazione. Nell'ultimo Consiglio dei ministri, quello di giovedì scorso, è stato approvato un decreto che ripristina le norme sull'espulsione dei clandestini; quelle norme che varie sentenze della magistratura avevano, di fatto, abrogato. Questo, infatti, è successo. L'anno scorso, la Corte costituzionale ha tolto l'aggravante al reato di clandestinità, che noi avevamo introdotto. Alcuni mesi dopo, sempre la Consulta, ha dichiarato che i clandestini, se in stato di indigenza, non possono essere espulsi. Poi, la Cassazione è intervenuta con altre sentenze. Hanno fatto di tutto per boicottare le nostre leggi sull'immigrazione! se ci sarà da fare una riforma della giustizia, la si dovrà fare per chiarire che il Parlamento fa le leggi e che i magistrati le devono solo applicare, non le possono cancellare.

Torna la linea del rigore e della fermezza, me lo lasci dire, signor Presidente, alla faccia di Vendola e della sinistra, che ci hanno attaccato per i contenuti di questo decreto. D'Alema si è detto indignato per le norme che abbiamo introdotto. Caro D'Alema, indignati pure, chi se ne frega: noi non vogliamo farci invadere dai clandestini, questo è il messaggio che vogliamo dare con forza sul territorio. Nel decreto abbiamo chiarito che l'unico posto dove possono stare i clandestini in questo Pese è all'interno dei CIE, reclusi all'interno dei CIE per essere identificati e poi espulsi. Noi sulle nostre strade non li vogliamo! I nostri Ministri stanno dunque lavorando al meglio, e adesso spetterà a noi parlamentari dare le risposte che i cittadini si attendono dalla nostra maggioranza. Come Capogruppo della Lega Nord, vi posso assicurare che ci impegneremo tutti al massimo, siamo già tutti pronti, tutto il Gruppo della Lega al Senato è pronto a lavorare per portare a casa risultati concreti nel più breve tempo possibile. Siamo Siamo anche tutti sull'attenti, agli ordini del nostro segretario federale Umberto Bossi: quello che ci dirà di fare, noi faremo.

E questo lo dico, signor Presidente, per rispondere a chi scrive sui giornali nazionali che la Lega è divisa. è divisa. I poteri forti hanno preso paura nel vedere la reazione del popolo della Lega a Pontida: questo è successo. Dopo i risultati delle ultime elezioni amministrative, pensavano e speravano in un clamoroso *flop*, ma così non è stato. Solo in pullman, sono arrivate a Pontida più di 80.000 persone, tutte con la camicia verde, tutte unite intorno ai vertici della Lega, ai nostri Ministri e a Umberto Bossi: questa è la Lega, e non è certo divisa. In tanti a Roma sognano una Lega divisa, ci hanno provato Lega divisa, ci hanno provato tante volte anche in passato e non ci sono mai riusciti, signor Presidente, perché noi abbiamo altro da fare che litigare, e questo lo voglio dire anche a chi è chiuso in qualche palazzo del potere in questo momento qui a Roma. Il nostro compito è molto chiaro: è quello di smantellare la struttura di questo Stato assistenzialista e centralista che ha prodotto negli anni il debito pubblico più alto in Europa e uno dei più alti nel mondo. È questo che vogliamo fare, ed è questo che faremo. *(Applausi dal Gruppo LNP).* Detto questo, abbiamo ascoltato attentamente, presidente Berlusconi, le sue parole, il suo intervento: molte delle nostre richieste sono state già accolte; affronteremo il problema del decentramento dei Ministeri in Parlamento, quando presenteremo la proposta di legge di iniziativa popolare. Oggi, dunque, confermiamo lealmente il sostegno a questo Governo, come abbiamo fatto in questi tre anni di legislatura: un sostegno al Governo, condizionato però, condizionato però, al rispetto dei tempi e all'approvazione delle norme e delle riforme che con forza il popolo della Lega ha richiesto a Pontida. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, l'assenza di contenuti nel suo intervento e anche il tono piatto con cui l'ha pronunciato ci confermano che non ha più niente da dire e da promettere all'Italia. La ripetizione è stanca, l'entusiasmo è spento, il messaggio è dimesso, e c'è da chiedersi se per primo ci creda lei.

un avanzo primario al 3 per cento (era a zero nel 2006), un debito pubblico decrescente, una procedura d'infrazione comunitaria revocata. Non sono lenti falsate a dirci che il nostro Paese oggi rischia il declassamento in ragione di un debito pubblico in aumento e di una crescita ferma; che la disuguaglianza è cresciuta penalizzando giovani, donne, il Sud del Paese (abbiamo i tassi di disoccupazione più alti d'Europa, e 2 milioni di ragazzi italiani non studiano, non lavorano, non si formano); che cresce l'iniquità stipendiale, pensionistica, fiscale; che l'Italia è sempre meno autorevole in campo internazionale; che la sua stessa persona è ragione di debolezza e non di forza nella relazione con altri Paesi. Ancora oggi, impegni internazionali già assunti diventano ostaggio di trattative politiche nel retrobottega del Governo. Il nostro è un Paese più vecchio e più chiuso. Si è fermato il processo di liberalizzazione, troppo sbrigativamente sostituito da privatizzazione di monopoli. Si è cercata forza nel consolidare privilegi e corporativismi, invece di aprire l'accesso alle opportunità economiche e alle nuove generazioni. La sfera pubblica è battuta e condizionata da personaggi che non hanno né titolo né responsabilità per determinare nomine e affari, attori di un'interlocuzione nella quale forte non è lo Stato né i suoi rappresentanti. L'intero impianto costituzionale è stato per anni, principalmente ad opera sua, signor Presidente del Consiglio, oggetto di attacchi tanto violenti quanto sconsiderati e inaccettabili. l'Italia intera ha subito e subisce una crisi economica grave che voi non avete determinato, ma alla quale non siete stati capaci di rispondere. Quel 13 maggio 2008 lei disse testualmente: «Crescere significa anche rilanciare il Paese e i suoi talenti, significa formare nuove generazioni di lavoratori altamente qualificati, significa dare una frustata vitale alla ricerca e all'istruzione». Se la frustata erano i tagli lineari del ministro Tremonti alla ricerca e all'istruzione e la riforma Gelmini, devo dirle che i giovani italiani, i docenti, le famiglie e il Paese intero hanno capito che quel termine non era usato metaforicamente. L'Italia non ha avuto nell'ultimo anno segnali di vitalità dal suo Governo: o fallimenti o immobilismi. Non esistono politiche industriali o del lavoro. L'ansia da prestazione del ministro Brunetta, piuttosto che esercitarsi su una riforma conclusiva e seria della pubblica amministrazione, si esaurisce nell'invettiva contro i soggetti che dovrebbe governare: in linguaggio calcistico, si direbbe un fallo da frustrazione. Il ministro Alfano ha sacrificato sull'altare della relazione politica con lei e con il PdL i suoi doveri costituzionali e la sua responsabilità. Il Piano per il Sud risulta ancora non pervenuto. Il federalismo che avevate promesso e sul quale, con lealtà e serietà di intendimenti e di proposte, ci avete incontrato, è nella sua attuazione roba buona per i comizi. L'hanno capito anche i sindaci leghisti, ai quali avete, nel frattempo, con la manovra economica e poi con il DEF, regalato due tagli da 16 miliardi ciascuno almeno, oltre al vincolo di stabilità per i comuni virtuosi, che ora volete abolire, o almeno dite di volere abolire,

dinanzi a Ministri della Repubblica che tacciono e coltivano l'ambiguità, indecisi se scendere da cavallo e cavalcare la tigre o mantenersi intanto intanto saldamente in sella sul destriero ministeriale. E nella notte, febbrili trattative per spostare Ministeri senza spostarli, per spendere di più senza spendere: una farsa, e anche una vergogna! Voglio dirlo chiaramente: quel 17 marzo, giorno dell'Unità d'Italia, non è stata una gloria breve, non ve la siete cavata - per quelli di voi che hanno partecipato L'unità è la ragione storica, politica e culturale dell'Italia. L'Italia c'è perché è unita, e la Repubblica è una e indivisibile;

Il 13 febbraio scorso per prime sono state le donne italiane, che hanno ancora raccolto e rilanciato la voce dei ragazzi e delle ragazze per l'istruzione, il sapere e il lavoro, che hanno mostrato proprio a lei, a migliaia in tutte le piazze italiane, di avere dell'Italia, e non solo di se stesse, un'idea dignitosa e fiera, e voi avete sbagliato assai a sottovalutarle. i risultati delle amministrative - avete perso le elezioni - e quindi i risultati dei *referendum*, che hanno in sé almeno tre significati. I cittadini non disertano le urne e rivogliono la parola;

Non dubiti, non siamo così sciocchi da pensare che quei voti siano nostri, anche perché il fatto più importante non è questo: a noi tocca il nostro lavoro, ma è più importante che il Paese sia sveglio e tutto in piedi, perché è questo il fatto politico. Veniamo a parlare della sua maggioranza: siamo qui per questo. Domenica, a Pontida, lei, signor Presidente del Consiglio, ha subito un'umiliazione molto grave. Ascoltavo Umberto Bossi, gli *slogan* degli intervenuti, il messaggio di quel raduno di popolo, e avvertivo il senso di quella che avrebbe dovuto essere la sua mortificazione (pensavo alla sua mortificazione): ma lei resiste anche a questo, e ciò purtroppo descrive l'abisso. Niente sarà più uguale. Ormai ad alzare la voce saranno autorizzati tutti. La sua maggioranza, ferita dallo strappo finiano, oggi è esposta ad ogni vento. Un pezzo importante ed autorevole dal punto di vista politico ed istituzionale l'ha abbandonata; ma nessuno riesce a rintracciare - noi siamo qui per questo - il senso e l'identità politica dei nuovi innesti della sua maggioranza, i Responsabili. Qualcuno sa che Italia vogliono, dove vogliono condurre il Paese, che programma politico hanno, fino a quando, e soprattutto perché votano, quando votano, appoggiando il Governo? È solo il partito del «portiamo a casa la legislatura» o è altro? E che cosa? Lei qui ostenta sicurezza, ma ormai credo che abbia il volo spezzato e breve di un calabrone che è finito dentro un barattolo di vetro. Lei, signor Presidente del Consiglio - il voto della Camera dei deputati oggi lo conferma - ha ancora la maggioranza, ipocrita, in Parlamento, ma fuori di qui, nel Paese, lei rappresenta la minoranza degli italiani. Non si affida ad un Presidente nelle sue condizioni, ad una maggioranza in queste condizioni, la guida di un grande Paese in difficoltà. Mi chiedo se lei sia davvero cieco e cosa aspetti: forse i pugnalatori nell'ombra, non lo so. Lei sta risultando il peggior carceriere di se stesso, ma insieme tiene in ostaggio Tre anni fa, con responsabilità, dicemmo che la crisi arrivava ed era seria, e voi spandevate ottimismo a buon mercato. Ora, con la stessa responsabilità, vi diciamo di andarvene. Democratico è probabilmente il primo partito italiano; sapremo saldare alleanze affidabili su un programma serio, cosa che voi non siete mai stati in grado neanche di pensare, oltre che di praticare. Noi sappiamo bene che le riforme strutturali di un Paese non possono farsi

credo che il discorso di oggi del Presidente del Consiglio sia stato importante per i contenuti, per i toni e per il modo con cui si è rivolto all'Assemblea del Senato e al Paese,

per la cassa integrazione, straordinaria e ordinaria, e le politiche del lavoro che voi avete contrastato. Cosa sarebbe oggi questo Paese se in anni passati non fossero state approvate leggi come la legge Biagi e norme sulla flessibilità? Cosa sarebbe stato questo Paese se governando voi a quei *referendum,* che qualche mese fa si sono tenuti a Pomigliano d'Arco o a Mirafiori e che hanno visto vincere lavoratori e sindacalisti coscienziosi, avesse vinto il no? Oggi staremmo a discutere dell'abbandono dell'Italia da parte della Fiat. Questa sarebbe la politica sociale e del lavoro che avreste realizzato. Quindi, credo che le cose dette oggi, le cose che conosciamo, i risultati anche della lotta all'evasione fiscale, che abbiamo condotto con cifre e con fatti, consentano al Governo di parlare di una delega per la riforma fiscale; di cui oggi il Presidente del Consiglio ha parlato con sobrietà, concretezza, scadenze e cifre. Una riforma fiscale che deve riguardare le famiglie, le imprese e il sistema produttivo. Tutto questo viene rivolgo ai colleghi dell'opposizione - avendo tenuto sotto controllo i conti pubblici ed avendo evitato all'Italia il collasso, pur in presenza di un debito così ingente vivendo altri Paesi; avendo evitato gli inasprimenti fiscali che hanno deciso gli inglesi o i licenziamenti in massa nel pubblico impiego che hanno attuato altri Paesi; e ancora, vi ricordate il film «Viva Zapatero» a cui inneggiavate? Zapatero in Spagna ha distrutto lo Stato sociale e portato al 20 Questa è la realtà dei numeri. Tutto questo in Italia non è avvenuto. C'è molto da fare, e la sfida di questo Governo è fronteggiare la crisi, ma affrontare anche la riforma fiscale, garantire lavoro e occupazione, prosciugare quelle sacche di precari che i Governi i Governi della sinistra hanno moltiplicato nella scuola e altrove, cari colleghi del Senato. *(Applausi dal Gruppo PdL).* È il pilastro dell'economia, del risanamento, dell'azzeramento del *deficit,* dei traguardi europei, della riforma fiscale e della sicurezza. chi, come il Governo Berlusconi, vara il codice antimafia, crea norme per arresti e sequestri di beni alle cosche, chi inasprisce il 41-*bis,* e chi nel passato quel carcere duro l'ha cancellato senza neanche chiedere scusa al Paese delle sue colpe e dei suoi misfatti. Siamo grati al presidente Berlusconi, al ministro Maroni, al ministro Alfano, che merita rispetto, come tutti gli altri, e scegliamo loro e il nostro Governo per la nostra fiducia. Voi avete scelto Ciancimino *junior* e le false icone dell'antimafia delle parole. Vergogna. Vergogna. Vergogna. Porteremo avanti la riforma costituzionale della giustizia, sulla quale chiediamo confronto e collaborazione. Garraffa. Richiami del Presidente)*. La lotta agli abusi di alcuni mezzi di indagine come le intercettazioni, la parità delle parti nei giudizi, la fine della politica tra le toghe, sono obiettivi importanti. Ma è tempo anche di riforme costituzionali, come ha ricordato oggi il presidente Berlusconi. Ricordo a coloro che, come noi, vogliono combattere i costi della politica, che se la sinistra, dopo un'effimera vittoria elettorale, non avesse spinto a votare in un *referendum* contro la riforma costituzionale che noi attuammo, oggi - nel 2011 - sarebbe già scattata la riduzione dei parlamentari. Noi realizzammo quella riforma: è inutile che voi, che la contrastaste con il *referendum,* riproponiate oggi questi temi. Noi vogliamo riprendere il cammino per una riforma del bicameralismo, per consentire ai cittadini piena scelta nell'elezione dell'Esecutivo e per una svolta presidenzialista che gli italiani auspicano. Vogliamo anche confrontarci sulla rappresentanza. Si discute molto delle leggi elettorali, ma sarebbe un paradosso se un *referendum* di cui si parla, per consentire al cittadino di scegliere tra un candidato e l'altro, realizzasse l'assurdo obiettivo di privare i cittadini della scelta del Governo, della maggioranza, del programma e del leader. Noi diciamo no a queste false riforme, perché vogliamo che i cittadini possano scegliere con il voto chi li governa e su quale programma deve governarli. Questo sarà un impegno prioritario per noi. Non vogliamo tornare indietro, al passato, quando il cittadino affidava la propria delega ai partiti, senza sapere che uso avrebbero fatto del suo voto: prima mi voti e poi ti dico con chi mi alleo. Diciamo quindi no a chi vuole scardinare il bipolarismo e tornare ai Governi fatti

- non vogliamo che si formino ammucchiate, ma aree programmatiche, fondate su valori comuni. Anni fa la sinistra vinse alcune elezioni amministrative e allestì la nota macchina da guerra, e ricordiamo tutti come andò a finire. Successivamente ci avete riprovato: tanti numeri, tante facce, Governi di oltre 100 membri (a proposito di costi della politica). Ci ricordiamo come è finita, perché non avete avuto nessuna omogeneità di programma. Vogliamo unire forze e ambienti nel quadro dei valori cui fa riferimento il Partito popolare europeo, di cui il Popolo della Libertà fa orgogliosamente parte. La politica di rinnovamento avviata all'interno del Popolo della Libertà guarda a questi obiettivi e traguardi con sincera apertura. Non vorremmo che qualcuno, in un polo, restasse spettatore inerte e passivo e diventasse strumento di una sinistra che, grazie alla passività di alcuni, potrebbe imporre valori sbagliati alla società italiana. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Riflettete, anche in altri settori del Parlamento, Siamo disposti al confronto per un incontro di aree omogenee che sia fondato su comuni scelte programmatiche e valoriali: non dimentichiamo le battaglie fatte in quest'Aula del Senato per difendere il diritto alla vita. Vogliamo unire su ciò che conta, e non tentare di sommare numeri che alle prime verifiche verrebbero cancellati dalla forza dei fatti. Sulla politica estera, a proposito di credibilità, l'altro giorno è venuto in Italia il *premier* di Israele Netanyahu, che ha dato atto al Governo italiano e al presidente Berlusconi dell'impegno in Medio Oriente - come ovunque - per difendere i diritti e le libertà, ambiguità e ammiccamenti a fondamentalismi di ogni tipo. *(Applausi dal Gruppo PdL).*Questo Governo ha garantito valori di libertà e di democrazia. Abbiamo dialogato con il Nord Africa. A proposito di missioni miliari, abbiamo visto che, sulla Libia, la sinistra si è scoperta interventista: avete messo dentro i cassetti le bandiere della pace, perché il vostro interventismo è solo strumentale per una politica di carattere interno e una polemica contro il nostro Governo. *(Applausi Un Governo che aveva espresso dubbi su alcune operazioni: fu il presidente Berlusconi (anche criticato per questo), ma la sua saggezza lo portava a vedere come era complesso quel quadro. Non ci siamo tuttavia sottratti ai nostri doveri di appartenenza alla coalizione internazionale, ma oggi è proprio il Governo Berlusconi - è stato detto quest'oggi - che rilancia iniziative politiche e diplomatiche perché si possa riportare pace e democrazia in Libia e in tutto il Mediterraneo. il Mediterraneo. Qualcuno aveva visto giusto, e nei giorni scorsi anche il Congresso americano ha dato dei voti che hanno espresso qualche dubbio. Anche in politica estera l'Italia, con il Governo Berlusconi, ha rispettato i propri impegni e confermato la solidarietà occidentale. Nelle aree più difficili di crisi del Medio Oriente e dell'Africa ha dimostrato la sua saggezza e utilità, e mette a disposizione questo patrimonio per tutto il Paese. Qualcuno pensava che oggi non avremmo più avuto di fronte a noi questo Governo; invece il Governo c'è, ha volontà di agire con rapidità e concretezza, ha consensi nel Parlamento, alla Camera e anche al Senato. Potevate presentare una mozione di sfiducia, se eravate così convinti che il Governo è delegittimato. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Non avete avuto la volontà di farlo; non avete avuto la forza di farlo. farlo. Mi consenta, Presidente, di ringraziare i senatori del Popolo della Libertà, e tutti i senatori della maggioranza, che hanno scelto la via della coesione e non quella della divisione, per il bene dell'Italia e per il sostegno a un Governo, che ha fatto l'interesse dell'Italia. Non ci sono alternative credibili a questo Governo, che deve andare avanti per attuare il programma che gli elettori hanno scelto con il loro voto. Lo abbiamo fatto in questi anni; continueremo a farlo per il bene dell'Italia e degli italiani.

Signor Presidente, ho chiesto la parola a fine seduta solo per evidenziare un aspetto di cui si è parlato molto in questi giorni, ossia la famosa questione del Patto di stabilità per i Comuni. Volevo ricordare ai colleghi parlamentari che su questo argomento è stato presentato un disegno di legge nel lontano ottobre 2008 che affronta la questione dei Comuni virtuosi e dei Comuni spreconi. Purtroppo, questo Parlamento non ha ancora affrontato tale argomento, e spesso e volentieri colleghi anche presenti qui stasera hanno preferito parlarne fuori, nelle piazze. Credo che il Parlamento debba ricondursi a quello che è il suo compito e il suo dovere, ossia risolvere le questioni e i problemi, e non strumentalizzarli. Pertanto, chiedo di portare attenzione a questa proposta e a quelle che sono quelle che sono state presentate da altri colleghi, proprio perché c'è assolutamente la necessità di dare risposta ai Comuni italiani, che spesso immaginano che in Parlamento ci siano dei marziani, visto che le norme che avete che avete approvato sul Patto di stabilità sembrano effettivamente fatte da persone che vivono al di fuori della realtà. *(Applausi